L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Compagnone e Arrigoni andremo ad illustrare. Va detto, a onor del vero, che avremmo gradito una discussione più ampia, con maggior tempo a disposizione dei vari Gruppi, anche perché

l'avvio della necessità del *decommissioning* dei quattro impianti nucleari esistenti nel nostro territorio e con l'indispensabile lavoro per la trattazione dei rifiuti nucleari e radioattivi esistenti, anche provenienti da attività industriali

che hanno collaborato alle relazioni e al lavoro svolto per queste quattro attività: l'ingegnere Mezzanotte, per quanto riguarda la mia relazione, e i magistrati Battarino

la criticità fondamentale; ovverosia, come è intuibile, l'assenza ad oggi di un deposito nazionale ove poter collocare i rifiuti radioattivi, distribuiti in vari punti del territorio nazionale, in massima parte laddove prodotti. Questa mancanza non consente una messa in stabile sicurezza dei rifiuti secondo gli *standard* oggi disponibili, rende incerta la prospettiva per le operazioni di *decommissioning* degli impianti nucleari e lascia irrisolta la questione dei rifiuti prodotti nell'impiego delle materie radioattive nella ricerca, nella sanità e nell'industria.

La seconda criticità che abbiamo evidenziato è la lentezza con la quale sono state condotte le attività di *decommissioning*. Ritardi già in partenza. Avrete modo di leggere nella relazione come si sia prolungato, quasi *sine die*, il tempo per il loro abbattimento e la loro trasformazione. Ma hanno contributo mutamenti di indirizzo politico per le scelte fondamentali, come per la gestione del combustibile irraggiato residuo. Ha contribuito l'inerzia, la farraginosità del complessivo sistema amministrativo e dei controlli. Ha contributo la ricordata mancanza di un deposito finale e l'obiettiva difficoltà e complessità delle operazioni da compiere. *(Brusio).* PRESIDENTE. Colleghi, vi invito ancora una volta a consentire alla relatrice di svolgere la relazione su un tema così delicato in condizioni idonee. Vi pregherei

nucleari dismessi, nonché di tutti i rifiuti radioattivi in Italia. Non ci sono solo cause endogene, ma anche cause tutte interne alla Sogin. Vi è un'ammissione, che si è avuta nell'ultima audizione dell'amministratore delegato Casale, il quale ha affermato come la mentalità prevalente all'interno della società sia quella di una gestione in sicurezza e dunque certamente positiva dal punto di vista della tutela dei lavoratori e dell'ambiente circostante, ma meno capace, meno propensa capace, meno propensa ad una programmazione complessa e specialistica, con le tempistiche ravvicinate, rigide e determinate che necessitano di un coordinamento e di una visione generale. La terza difficoltà che evidenziamo riguarda le funzioni di controllo ed è una difficoltà alla quale il Governo deve davvero porre immediato rimedio. Funzioni che sono state attribuite nel 1994 ad ISPRA,

Con l'ultimo decreto n. 45, in relazione all'attuazione della direttiva EURATOM 70 del 2011 in materia di gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, è stato istituito l'ISIN, l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione. È prevista una struttura di almeno 60 tecnici, in particolar modo ingegneri nucleari specializzati; ma né la dirigenza né la struttura sono mai state attivate. La Commissione rileva la vetustà degli attuali tecnici presenti in ISPRA, tutti *over* 50 e la situazione del dimezzamento, determinato da quiescenze.

ammettere che la comparazione con le altre realtà internazionali - la Francia e la Spagna - rende ancora più chiaro, da una parte, il cammino che dobbiamo fare e, dall'altra, le evidenti

ma proprio questo non deve portarci sulla cattiva strada di ritenere che sia banale ciò che stiamo facendo: non lo è per nulla. La dimostrazione - come vi dicevo - sta proprio nella preoccupazione che cresce negli ambiti territoriali in cui sono attualmente i sistemi e gli impianti in forma provvisoria. Cosa sta accadendo in Spagna, molto più simile a noi in relazione al tema della trattazione dei rifiuti radioattivi? Siamo andati a Cordoba, ad El Cabril, nella provincia andalusa, e abbiamo verificato che un impianto superficiale di smaltimento dei rifiuti a bassa e media attività, molto simile al nostro per caratteristiche strutturali e modalità di gestione, è stato già realizzato. Ebbene, è quasi incredibile, sapendo ciò che accade nel nostro Paese, apprendere che quell'impianto gode di un altissimo livello di sicurezza e della complessiva serenità di tutta la popolazione che vi vive accanto. Va detto che, proprio recentemente, un bando per la partecipazione

Questo ci permette di dire, proprio trasferendo le informazioni ricevute, che per permettere gli insediamenti nazionali di stoccaggio dei rifiuti nucleari è necessario un cambio di marcia che veda totale trasparenza nelle informazioni e nelle procedure, una partecipazione attiva della popolazione, la credibilità dei gestori e dei controllori, la chiarezza da parte dei Governi. Da agosto attendiamo l'autorizzazione alla Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee per proseguire questo cammino, per mantenere gli impegni internazionali che abbiamo assunto e per dare garanzia e conferma alle popolazioni italiane che questo Governo e questo Parlamento stanno facendo sul serio. C'è il rischio che si apra un'infrazione comunitaria per non aver ottemperato nei tempi previsti alla creazione della Carta dei rischi e all'individuazione e alla realizzazione del deposito nazionale. Sottolineo, quindi,

n. 8*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, sottosegretario Degani, l'attività d'indagine sulla Liguria ha avuto inizio con una missione svolta dal 20 al 23 gennaio 2015. Si è preceduto all'audizione di autorità giudiziarie, autorità amministrative, associazioni ambientaliste e rappresentanti sindacali, nonché all'effettuazione di numerosi sopralluoghi presso il porto di La Spezia, il sito di Pitelli, la discarica di Genova-Scarpino, il porto di Genova dove allora si trovava L'indagine conoscitiva proseguiva con una seconda missione a Genova e ad Imperia dal 18 al 20 febbraio 2015. Un *focus* è stato realizzato sull'Agenzia delle dogane e sul traffico transfrontaliero dei rifiuti, con ispezione nelle sedi di movimentazione dei *container*. È stato svolto un sopralluogo al SIN di Cogoleto, in Provincia di Genova, e una visita presso la discarica di Collette Ozotto a Taggia, in Provincia di Imperia. Sono stati complessivamente acquisiti 113 documenti provenienti da soggetti pubblici e privati. Per comprendere quanto è avvenuto nella Regione Liguria non si può prescindere dalle sue peculiarità: una Regione con 330 chilometri di costa,

per densità abitativa in Italia. A questa forte concentrazione di popolazione si associa, peraltro, un tessuto produttivo notevole con grandi porti (Genova, La Spezia: i due porti più grandi in Italia), attività turistico-commerciali, attività artigianali sviluppate, grandi poli industriali per la raffinazione del petrolio, la cantieristica navale e la produzione di energia. Tutto questo in una Regione con un territorio piccolo, come abbiamo detto, prevalentemente montuoso che declina direttamente sul mare. Un'altra nota importante è che vi è una produzione *pro-capite* di rifiuti di ben il 14 per cento in più rispetto alla media nazionale. Quindi, una Regione con particolari caratteristiche orografiche, altamente urbanizzata, dove insistono porti e attività industriali, avrebbe dovuto dotarsi di una strategia adeguata per la gestione sostenibile dei rifiuti. Questo non è avvenuto; nel tempo si è ipotizzata la realizzazione di strutture tecnologicamente avanzate e straordinarie che avrebbero dovuto risolvere i problemi, ma in realtà non sono mai state realizzate, lasciando esposto il territorio ad una *deregulation* con fenomeni di illiceità, solo in parte scoperti e comunque sempre da temere. Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti urbani, la Regione ha basato tutto sulla presenza di ben 174 siti di discarica distribuiti nelle quattro Province, dei quali solo 52 sono stati dichiarati definitivamente bonificati solo due sono attualmente funzionanti (Collette Ozotto e Rio Marsiglia) per un progressivo ed ineluttabile esaurimento della capienza di tutti gli altri siti. Pertanto, questo sistema fortemente dipendente dagli impianti di discarica è entrato inevitabilmente in crisi, con la conseguenza che una grande quantità di rifiuti viene esportata fuori Regione per lo smaltimento in base ad accordi interregionali. Tutte le altre forme di gestione appaiono residuali, tant'è che i livelli di raccolta differenziata si attestano intorno al 30-33 per cento. Esistono solo 5 impianti di compostaggio in tutta la Regione che hanno trattato nel 2013 soltanto 24 tonnellate di rifiuto organico, quindi il recupero della frazione organica si attesta a quote veramente modeste. In Liguria, peraltro, non è presente alcun impianto di digestione anaerobica. Il trattamento meccanico biologico utilizzato unicamente come forma di pretrattamento dei rifiuti da avviare in discarica conta solo due impianti. Pertanto, oltre i due terzi dei rifiuti collocati in discarica non è sottoposto ad alcuna forma di pretrattamento come la normativa vigente, specie Non esiste, tra l'altro, alcun impianto di valorizzazione energetica del rifiuto. Per quanto riguarda i rifiuti speciali, in Liguria esistono - ribadiamo - poli industriali importanti per cui si riscontra una notevole produzione di rifiuti chimici e siderurgici, nonché produzione di rifiuti derivante dall'attività portuale, del settore navale della produzione di energia elettrica. A questi vanno aggiunti i rifiuti inerti da costruzione e demolizione, i rifiuti di amianto e quelli derivanti da terre e rocce da scavo. Tale tipologia di rifiuti rappresenta un punto sensibile per questa Regione, considerando sopratutto le grandi opere in corso Si tratta di enormi quantità: quasi 16 milioni di metri cubi di terre e rocce da scavo utilizzati come sottoprodotti e due milioni di metri cubi gestiti come rifiuti. Liguria sono sostanzialmente due: da un lato, la carenza di impiantistica adeguata; dall'altro, la mancanza di una *governance* efficace e di una strategia complessiva della gestione dei rifiuti. I soggetti gestori sono parecchie decine, frammentati sul territorio, con situazioni miste e manifestano una inadeguatezza generale del sistema. La situazione che grava oggi sulla città metropolitana di Genova e sulla Regione è quella di un ritardo grave nel perseguimento degli obiettivi di differenziata e di un persistente sistema diseconomico ambientalmente negativo, basato sul trasferimento dei rifiuti. Tutto questo comporta chiaramente un possibile terreno di coltura di forme di illegalità diffusa e di infiltrazioni criminali, più o meno organizzate. Nel gennaio 2015 è stato presentato in Commissione bicamerale il nuovo Piano di gestione dei rifiuti, successivamente integrato e approvato nel marzo 2015 e notificato al Ministero. Questo Piano è basato sull'individuazione dell'ambito regionale unico, articolato in aree territoriali corrispondenti al territorio della città metropolitana di Genova e delle tre Province di Imperia, Savona e La Spezia. Esso contiene indirizzi e strategie per la gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali e le operazioni di bonifica da attuarsi entro il 2020, indicando le modalità di una evoluzione complessiva del sistema verso gli obiettivi previsti a livello comunitario e nazionale. Esso individua inoltre la Regione come autorità d'ambito per il governo del ciclo dei rifiuti, attraverso un comitato d'ambito costituito dal presidente della Giunta regionale, dal sindaco della città metropolitana e dai presidenti delle Province, demandando la più

Gli impianti per la depurazione delle acque reflue urbane rispecchiano la distribuzione della popolazione: vi sono grandi impianti nelle zone costiere e piccoli impianti nell'entroterra. Più di un terzo di questi difetta di conformità alla normativa; impianti non adeguati, ma autorizzati nelle more dell'adeguamento, mentre altri adeguati sono in attesa di autorizzazione. La Liguria si affaccia sul mare con i due grandi porti di Genova e La Spezia, che - come sappiamo - sono tra i porti più grandi d'Italia; un terzo porto è quello di Savona. Tali porti, avendo alle spalle tutta la zona padano-alpina, con le grandi realtà produttive del Nord, costituiscono un territorio particolarmente sensibile ai traffici internazionali, anche di natura illecita. Tra le autorità che forniscono attività di contrasto alle attività illecite in area portuale (Capitanerie di Porto e Agenzia delle dogane) e le polizie giudiziarie, nonché le procure della Repubblica, si è riscontrata da parte della Commissione una collaborazione effettiva effettiva ed efficace, che ha permesso di evidenziare le dimensioni rilevanti e in crescita del fenomeno del traffico transfrontaliero dei rifiuti; un vero e proprio fenomeno di *dumping* ambientale, ad opera di soggetti spesso stranieri, con la correità di intermediari italiani, che porta ad eludere le norme italiane sui rifiuti, organizzandone il trasferimento all'estero, laddove discipline più permissive o meno capaci di controllo diventano la sede utile ove svolgere attività di sfruttamento del rifiuto attraverso modalità altamente inquinanti, con il finale abbandono incontrollato dei residui. Tutto ciò ha un impatto negativo sul circuito economico nazionale, poiché all'economia del nostro Paese viene sottratta una ingente quantità di materia da destinare al riciclo e al riuso. due grandi criticità in questo meccanismo di contrasto al traffico transfrontaliero. Anzitutto c'è una quantità enorme di materie che passa anche per altre vie, oltre che per i porti; essa arriva soprattutto dai Balcani, su gomma ad esempio, sfuggendo ai normali controlli.

conclusione mi corre certamente l'obbligo di ringraziare i funzionari della Commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, in particolare il dottor Battarino, che è stato un ottimo e straordinario collaboratore. Ringrazio altresì il nostro presidente, Alessandro Bratti, tutti i colleghi parlamentari e soprattutto il collega Mario Morgoni, che con me ha relazionato sulla Liguria e si è occupato

trasparenza e dunque consapevolezza da parte di voi colleghi rispetto ad alcune situazioni, anche gravi, complesse e problematiche, presenti sul territorio nazionale. Il contingentamento dei tempi tantomeno potrà consentire ragionamenti generali sul futuro della chimica del nostro Paese, un settore industriale grande protagonista del passato, che esattamente cento anni fa, nel 1916, aveva dato vita alla prima forma di associazionismo tra le imprese. Penso ad esempio agli interrogativi su quale sarà l'impegno futuro di ENI nella chimica. Ma tant'è: proseguiamo. La Commissione, che ha iniziato la propria attività nel settembre 2014, sta facendo approfondimenti a carattere territoriale,

di non procedere - come fatto in passato - con un'unica relazione ricognitiva, che vedrebbe la luce solo a fine legislatura, ma di preferire l'esame dei singoli siti più importanti mediante appositi approfondimenti. È questo il caso della situazione di cui discuteremo oggi relativamente al sito di interesse nazionale di Porto Marghera e quella successiva del cosiddetto quadrilatero della chimica. La relazione sulla bonifica del SIN di Porto Marghera è stata approvata all'unanimità dalla Commissione lo scorso 10 dicembre 2015. Il sito di Marghera fa parte, dal punto di vista produttivo, dell'importante quadrilatero della chimica. Marghera è stato sicuramente uno dei siti industriali più importanti del Paese per quanto riguarda la chimica. L'industria chimica, come è noto, in quanto radice di ogni altra, se da un lato è stata alla base dello sviluppo di tutta l'industria

e comprendeva oltre 3.200 ettari di aree di terra, 350 ettari di canali portuali e interessava 2.200 ettari di area lagunare; oggi il SIN, in base a tutta una serie di interventi e di riperimetrazioni, è di circa 1.620 ettari. Lo spettro impattante dei contaminanti trovati è frutto di un'eredità industriale e del modo di produrre in passato: nei suoli sono state trovate varie tipologie di metalli, così come nelle acque di falda, dove, oltre ai metalli, sono stati rinvenuti anche idrocarburi policiclici aromatici. Si tratta, dunque, di un processo di inquinamento molto forte, che ha visto impegnati fin dal 1998 diversi enti nel tentativo di mettere in sicurezza e bonificare Ad un primo accordo di programma del 1998 è seguito nel 2004 un *masterplan* che coinvolgeva un po' tutti gli attori istituzionali e che prevedeva la messa in sicurezza permanente di Porto Marghera; successivamente sono stati redatti altri accordi di programma, tra cui quello significativo del 2012 e l'ultimo del 2015. Tra i vari accordi è significativo quello del 2006 che faceva riferimento al magistrato delle acque di Venezia e al proprio concessionario, il Consorzio Venezia Nuova, proprio quello noto alla triste cronaca per le questioni legate ai lavori del MOSE; questioni non indipendenti, ma anzi fortemente intrecciate a quelle della bonifica del sito di Porto Marghera. Come Commissione abbiamo innanzitutto

Per quanto riguarda la messa in sicurezza delle macroisole, che suddividono quest'area molto vasta mediante la posa in opera di palancole che realizzano i cosiddetti marginamenti atti ad impedire agli inquinanti di uscire in laguna, ad oggi lo Stato ha sostenuto una spesa complessiva di oltre 780 milioni di euro, di cui, come detto, più di 500 derivano dalle transazioni fatte con le imprese che più hanno inquinato. Di fatto, in termini di lunghezza dei marginamenti, è stato realizzato il 94 per cento delle opere previste. Ne risultano ancora da eseguire circa 3,5 chilometri, corrispondenti al 5-6 Quello che rileva, purtroppo, è che per realizzare quella che, ad una lettura sommaria, sembrerebbe una parte residuale delle opere mancanti servono in realtà altri circa 250 milioni di euro di risorse statali, un importo sproporzionato rispetto a quanto speso, ma giustificato dal fatto dal fatto che mancano (anzi, sono state lasciate per ultime) proprio tutte le aree più complesse, ad esempio quelle dove passano le sottostazioni. In sostanza, siamo di fronte ad opere di marginamento imponenti ma che presentano diversi varchi che, allo stato attuale, vanificano l'obiettivo di isolare queste isole della laguna. A seguito di quanto realizzato, che simbolicamente potremmo definire un colabrodo, gli inquinanti di fatto continuano ad uscire e il sistema drenante diventa assolutamente inefficiente ed inefficace. Significativa in merito in merito è una dichiarazione, che definirei imbarazzante, da parte dell'attuale Provveditore per le opere pubbliche, audito dalla Commissione, che ha parlato di mancato controllo delle opere realizzate. In realtà, i lavori sono stati assegnati senza gara ad evidenza pubblica, in barba a qualsiasi tipo di normativa italiana e non vi sono stati neanche una verifica e un controllo sullo stato dei lavori. Come Commissione con viva preoccupazione abbiamo segnalato questa assurda e delicata situazione che, inevitabilmente, deve chiamare tutti ad un senso di responsabilità. Questo a prescindere dalle colpe di chi non ha realizzato in maniera adeguata quell'opera, perché il rischio che continui l'inquinamento e soprattutto che si possa riaprire il contenzioso tra lo Stato e le imprese che hanno pagato, attraverso le transanzioni, il corrispettivo per addivenire all'emergenza delle bonifiche è molto è molto forte. Ad oggi i fondi a disposizione sono assolutamente insufficienti per terminare quell'opera. Infatti, attraverso le rate delle transazioni già firmate con le diverse imprese, che terminano circa nel 2023, si ipotizza possano giungere al massimo 30 milioni di euro, ben lontani dai 250 necessari. necessari. La mancata bonifica e messa in sicurezza di Porto Marghera rappresenta un serio ostacolo per un processo per di reindustrializzazione di quell'area, che peraltro presenta tante manifestazioni di interesse da parte dei privati.

assegnati attraverso decine di commissioni a funzionari ministeriali e locali che hanno collaudato a pezzi l'opera, senza mai pervenire ad un collaudo generale e definitivo. Si tratta, ad avviso della Commissione, di 2 milioni di euro spesi molto male. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo in breve sintesi è il lavoro che è stato portato avanti dalla Commissione e che oggi è a disposizione delle diverse forze politiche per le opportune considerazioni. Ora auspichiamo, visto che è l'obiettivo che ci siamo dati come Commissione, che queste denunce, anche attraverso l'approvazione di una risoluzione, si trasformino per chi di dovere *in primis* il Governo - in atti concreti per cercare di risolvere il problema denunciato. Non si tratta solo di salvaguardare il lavoro fatto sui marginamenti,

vorrei sottolineare che tutti i Gruppi politici hanno collaborato positivamente per giungere ai risultati in essa contenuti. Inoltre, vorrei soprattutto ringraziare le persone che hanno reso possibile il lavoro è stato svolto, dunque tutti gli uffici, i consulenti, i rappresentanti delle Forze dell'ordine e, soprattutto, il dottor Castellano e il dottor Battarino, i due magistrati che sono stati un punto di riferimento della presente relazione e di quella sul Quadrilatero, che mi

febbraio, emerge chiaramente che la messa in sicurezza e la bonifica dei siti industriali contaminati comportano un'impellente necessità di intervento, sia per l'esigenza di eliminare le fonti di inquinamento nei suoli, nei sottosuoli, nelle acque superficiali e nelle falde, al fine di garantire la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, sia per permettere la reindustrializzazione di aree strategicamente posizionate e adeguatamente asservite da infrastrutture, così da assicurare lo sviluppo industriale del Paese, difendendo contemporaneamente l'esigenza di evitare l'ulteriore Il cosiddetto Quadrilatero del Nord dell'industria chimica, formato dai poli di Venezia, Porto Marghera, Mantova, Ferrara e Ravenna, ha rappresentato dagli inizi del Novecento - lo ripeto - la storia

un inquinamento ambientale consistente che occorre risolvere nel migliore dei modi e con urgenza. La relazione specifica della Commissione espone le diverse metodologie di approccio adottate dal Governo e dagli enti territoriali per la gestione della bonifica dei singoli siti, con lo scopo - si spera - di orientare le scelte del Governo e del Parlamento verso la risoluzione più efficace delle criticità riscontrate. Lo sgravarsi di responsabilità tra gli enti pubblici coinvolti, l'assoluta complessità e frammentarietà della normativa in tema di bonifiche, le accuse reciproche tra il comparto il comparto pubblico e quello privato sui tempi, sui limiti restrittivi e sulle difficoltà dei controlli hanno spesso intralciato le operazioni di bonifica e i procedimenti amministrativi per sfociare in interminabili procedimenti giudiziari che hanno bloccato le attività. Sottolineo che non si registrano solo tecniche dilatorie intraprese da aziende coinvolte nei processi di bonifica che impugnano davanti al TAR i provvedimenti della pubblica amministrazione o anche quelli usciti dalle Conferenze dei servizi, con con lo scopo di evitare gli investimenti necessari in base alle prescrizioni impartite. Spesso dalla parte privata il contenzioso amministrativo è inteso - a volte a ragione - quale forma di tutela resa necessaria da prescrizioni ritenute inattuabili, irragionevoli o anche o anche soltanto derivanti da inadeguatezze tecniche dei tavoli o da conduzione tecnico-giuridica inadeguata delle Conferenze e dei rapporti tra le parti. Siamo certi che l'introduzione tra i reati ambientali del codice penale del reato di omessa bonifica costituirà una leva importante in mano alla magistratura per far maggiormente rispettare i procedimenti in atto di messa in sicurezza e di bonifica. Indubbiamente, fino ad oggi è stata la carenza di risorse il maggior ostacolo alla conclusione delle attività di bonifica. È stato riscontrato che, laddove nei siti permane l'interesse privato per la prosecuzione delle attività industriali, con annesso impegno finanziario privato, le attività di bonifica procedono con risultati positivi, mentre rallentano sino a bloccarsi nel caso contrario, a causa della carenza di risorse pubbliche. I due esempi/modelli di bonifica dei siti di Ferrara e Ravenna, che non sono siti di importanza nazionale e rientrano nell'esclusiva competenza regionale e locale, hanno hanno dimostrato l'importanza di organizzare un'interlocuzione efficace tra le industrie private attive nel sito e l'amministrazione pubblica, attraverso accordi di programma, e hanno comprovato la grande importanza che può avere il dialogo costruttivo tra le parti e la riduzione del numero e della distanza dal territorio degli interlocutori pubblici; a ciò si aggiunge l'imprescindibile necessità della permanenza delle attività industriali nei siti e della prospettiva del riuso delle aree per attività produttive. In questi due siti di interesse regionale, con gli accordi di programma tra enti locali e imprese, le bonifiche sono procedute a dei livelli soddisfacenti, perché in entrambi i casi le imprese hanno costituito un organismo unico che fa da interlocutore con la parte pubblica, cioè Regione ed enti locali. Al contrario, le attività di bonifica del SIN di Venezia-Porto Marghera (l'altro modello) hanno fatto emergere tutte le carenze e distorsioni dell'elefantiaco sistema burocratico-amministrativo centralizzato, con sperpero di risorse pubbliche, irregolarità nell'assegnazione degli appalti e cattiva organizzazione degli investimenti. Certo, Porto Marghera è una realtà molto diversa da quella dei due siti di Ferrara e Ravenna, in particolare per l'estensione dell'area inquinata e per la peculiarità delle caratteristiche del sito lagunare. Ma il problema più evidente - certamente connesso all'illogica ed inefficace parcellizzazione nell'esecuzione delle opere di marginamento (e rifacimento delle sponde delle macroisole lagunari) suddivisa tra il Provveditorato, la Regione Veneto e l'Autorità portuale, pur essendo gli oneri economici a carico del Ministero dell'ambiente - è rappresentato dall'esigenza di un immediato ulteriore stanziamento di 250 milioni da parte del Governo per completare i marginamenti; diversamente, si rischierebbe l'indebolimento dei tratti terminali dei marginamenti già effettuati, con grave pregiudizio per il complesso delle opere che sino ad oggi hanno comportato, come ho detto, una spesa per lo Stato di circa 780 milioni di euro. euro. Il SIN Laghi di Mantova e Polo chimico ha invece evidenziato una realtà molto composita, con una pluralità di soggetti privati che spesso non si raccordano tra loro, con progetti e una pluralità di interventi di soggetti pubblici aventi ruoli asimmetrici e difficoltà di organizzare un'interlocuzione efficace e non conflittuale tra l'amministrazione pubblica e i soggetti privati coinvolti. Tale situazione ha generato una serie di contenziosi giudiziari che

Grazie dell'amministrazione pubblica ed in particolare del Ministero dell'ambiente, con capacità di interlocuzione tecnica elevata e costruttiva con gli enti territoriali e con i soggetti privati. Inoltre, una questione che il Gruppo della Lega Nord e Autonomie ha più volte evidenziato e posto, anche con emendamenti specifici alla legge di stabilità (ahimè, respinti), e che è stata al Governo anche dalla Commissione d'inchiesta, è quella della necessità di prevedere l'esclusione dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica delle risorse destinate dagli enti locali alle bonifiche. Riteniamo che una tale previsione potrà costituire un sostegno concreto per le bonifiche di una serie di siti inquinati minori sparsi sul territorio che rappresentano problematiche importanti per le realtà territoriali e per la tutela della salute dei cittadini. Concludo, signor Presidente, con l'auspicio che la relazione della Commissione d'inchiesta possa servire da stimolo per il Governo per una gestione più efficace delle operazioni di bonifica dei SIN, ai fini della riconversione industriale delle aree del Paese e il rilancio del settore della chimica e della ricerca tecnologica nel nostro Paese. *(Applausi dei

Signor Presidente, inizio deprecando anch'io questo contingentamento dei tempi di discussione generale, perché ritengo sia veramente poco rispettoso delle minoranze. Non è questo il modo di procedere: troppo poco tempo per materie così importanti. Nugnes)*. La gestione e la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi è ancora un problema irrisolto. È un argomento talmente complicato che perfino il Governo Berlusconi inciampò nel 2003 davanti alla forza di una protesta pacifica, che durò 15 lunghi giorni contro l'imposizione di ubicare a Scanzano Jonico, in Basilicata, un deposito di scorie nucleari. Da allora sono passati molti anni ma ben poco è cambiato, nel senso che i rifiuti da gestire sono lì e sono gli stessi di sempre. I Governi che sono seguiti, per incapacità o mancanza di volontà, non hanno affrontato l'argomento per il quale si è ancora alla ricerca di soluzioni. Forse il tema per la politica è troppo impopolare e poco elettorale, quindi si preferisce spostare la patata bollente sempre più in là. Le conseguenze di questa indifferenza sono pericolose e costose. Pericolose per la salute dei cittadini che convivono con i centri nucleari, dato che secondo l'Istituto superiore di sanità sussistono, nei comuni sedi di impianti nucleari, alti tassi di decessi per patologie connesse all'esposizione a radiazioni ionizzanti. Ricordo che la suddetta ricerca dell'ISS ha riguardato la mortalità delle popolazioni residenti in otto cittadine italiane prospicienti a siti sede di attività di ricerca o a depositi di materiale radioattivo. Gli avvenimenti di Latina in questi ultimi giorni e quelli accaduti precedentemente negli altri centri dovrebbero farci capire quanto sia importante intervenire con urgenza. Invece, per irresponsabilità del Governo e per problemi interni alla *governance* di Sogin, più volte portati dal sottoscritto in 10a Commissione all'attenzione del Presidente e dei colleghi, continuiamo irresponsabilmente a rinviare le soluzioni, con un ritardo dei programmi di *decommissioning* che ha generato un aumento delle previsioni di spesa, spesa, passate dai complessivi 4,35 miliardi di euro stimati nel 2006 ai 6,7 miliardi stimati nel 2011, al netto dei costi della realizzazione del deposito nazionale, valutati in 1,5 miliardi di euro. costi posti a carico dei cittadini attraverso una specifica componente tariffaria (A2) nella bolletta elettrica, bolletta che peraltro aumenterà anche per la chiusura del mercato tutelato, una delle poche cose che funzionavano in Italia. Peccato. Come viene riportato nella risoluzione i programmi generali approvati nel 2013 dai nuovi organi della Sogin presentano, rispetto alla programmazione precedente, uno slittamento del termine degli smantellamenti che va da un minimo di due a un massimo di nove anni, a seconda del sito nucleare cui si fa riferimento. L'allungamento dei tempi è determinato da una serie di inadempienze interne al processo dell'attività di messa in sicurezza, delle quali, per mancanza di tempo, Vi è l'inadeguatezza della struttura di controllo, attualmente in capo all'agenzia di protezione ambientale ISPRA: il dipartimento al quale sono affidati i compiti dell'autorità di sicurezza nucleare ha visto, nell'arco degli ultimi sei anni, più che dimezzarsi il personale tecnico di cui disponeva, pur rappresentando, ad oggi, le sole competenze nazionali esistenti in materia di regolamentazione e controllo delle attività nucleari. Questa carenza di personale proietta difficoltà anche sul futuro dell'ISIN, l'Ispettorato istituito dal decreto legislativo n. 45 del 2014 per svolgere le funzioni oggi affidate all'ISPRA, il quale dovrebbe avere, secondo la legge istitutiva, un organico di sessanta tecnici. Ma vi è un altro problema ancora più grave: l'istituzione dell'ISIN è bloccata dalla nomina del suo direttore, individuata dal Governo in Antonio Agostini secondo un criterio fiduciario. Agostini possiede un profilo professionale fortemente criticato per l'incompatibilità rispetto al ruolo che dovrebbe ricoprire e la mancanza delle competenze tecnico-scientifiche invece obbligatoriamente prescritte dalla direttiva comunitaria. Quindi, cari colleghi, questa nomina è bloccata con una responsabilità precisa del Presidente del Consiglio, che ha investito Agostini

richiede che ogni Stato membro predisponga e trasmetta alla Commissione europea, entro il 23 agosto 2015, un programma nazionale per la gestione del combustibile nucleare irraggiato e dei rifiuti radioattivi; Auspichiamo che tale programma venga messo al più presto in consultazione, fase nella quale è prevista la partecipazione e il coinvolgimento delle popolazioni interessate. Ulteriori ritardi rispetto alla definizione di tale indispensabile programma rischiano di far permanere questo stato di inadempimento sul problema, provocando tra l'altro l'apertura di una ennesima procedura di infrazione da parte della Commissione europea. Concludendo, signor Presidente, siamo curiosi di sapere se al *summit* di Washington sulla sicurezza nucleare il presidente del Consiglio Renzi illustrerà la situazione reale in cui versiamo, per cui ci troviamo di fronte ad un' Italia che non ha fatto i compiti prescritti ed è in stallo, proprio per la responsabilità del Governo Renzi, a causa della suddetta vicenda ISIN - il blocco per la nomina di Agostini - o se racconterà la solita favoletta per cui in Italia va tutto bene. Signor Presidente, anch'io vorrei preliminarmente ringraziare il collega Compagnone, i colleghi della Commissione Grazie La Commissione, nell'ambito dei propri lavori, ha esaminato le criticità sulle quali si sono concentrate le attività di polizia e di prevenzione, costituite fondamentalmente dalla movimentazione di rifiuti con altre Regioni, dalle attività di bonifica e dalla gestione dei materiali di scavo, come rocce e terre. In termini generali, possiamo dire che in questa Regione si assiste alla compresenza di tre fenomeni: una microillegalità piuttosto diffusa e uniforme, gli illeciti ambientali derivanti dalla gestione di impianti di grandi dimensioni e i rischi di permeabilità del sistema, soprattutto nelle società che si occupano di gestione dei rifiuti per conto dei Comuni. permeabilità è di carattere prevalentemente corruttivo e non legata alla criminalità organizzata. L'estrema frammentazione nella gestione dei rifiuti è stata già sottolineata: fino ad un paio di anni fa esistevano circa 40 operatori privati, che si occupavano della gestione dei rifiuti e oggi tale realtà è dimezzata. Questa frammentazione, che continua a caratterizzare il sistema della Liguria, rappresenta un punto di accesso per interessi illegali, così come un sistema incentrato sulle discariche, che in molti casi sopravvivono a se stesse, può diventare alimento di rilevanti interessi illeciti. In ogni caso, la parcellizzazione dei servizi ha anche un'ulteriore ricaduta negativa, in quanto non agevola certo l'attività di controllo da parte delle forze di polizia, perché questa pluralità e molteplicità di soggetti rende indubbiamente più difficoltosa l'attività di contrasto all'illegalità. Tutti questi fattori richiamano la necessità di una razionalizzazione della gestione, che deriva ovviamente da un'efficace pianificazione, ma anche da una concreta capacità di attuazione della stessa. Inoltre, il costante stato emergenziale che ha caratterizzato in questi anni la Liguria e gli elevati interessi economici finiscono per facilitare, in presenza di procedure spesso adottate in via d'urgenza, una gestione non del tutto trasparente degli appalti. Non si può parlare, in Liguria, di una presenza diffusa e pervasiva della criminalità organizzata nel settore dei rifiuti, ma indubbiamente vi sono tentativi di infiltrazione nel tessuto sociale ed economico, perpetrati in modo poco appariscente e cogliendo le occasioni che offre l'economia legale, come l'affidamento di appalti e subappalti di servizi, compresi quelli relativi allo smaltimento dei rifiuti. l'indagine "La svolta" ha rappresentato un preoccupante segnale per quanto riguarda la presenza della criminalità organizzata, sebbene su altri versanti e non su quello dei rifiuti. quella indagine è stata coinvolta, ad esempio, la famiglia Pellegrino, che aveva interessi nel settore del movimento terra, ovvero in un settore collegato agli scavi, che richiede un bassissimo *know-how* ed è strettamente legato al tema dei rifiuti, come dirò successivamente. Ad esempio Ad esempio nei lavori del Terzo valico dei Giovi vi sarà il conferimento di circa 5 o 6 milioni di metri cubi di materiale, in oltre una decina di siti, cave ed ex cave. Nel lavoro della Commissione è emersa la sollecitazione ad incrementare anche il controllo su strada del trasporto dei rifiuti, visto che chi trasporta rifiuti illegalmente opera in nero, senza iscrizione all'albo dei gestori ambientali e quindi senza poter accedere ad impianti di smaltimento e di recupero. In questo contesto problematico si evidenzia comunque una forte capacità di collaborazione

l'utilità di un ancor più stretto coordinamento tra i soggetti che hanno competenza di prevenzione e polizia giudiziaria nel settore. Vi sono esempi di buona prassi in Liguria in questo senso, ma forse occorrerebbe dare risposte più incisive con appositi interventi normativi a questa esigenza importante. Anche in Liguria la Commissione ha verificato la criticità costituita dall'attribuzione di competenze alle procure distrettuali del reato di cui all'articolo 260 del Testo unico ambientale. Ovviamente, la materia è controversa, ma prevale un giudizio negativo su questa attribuzione, in quanto c'è una privazione delle procure territoriali della possibilità di agire e intervenire su fatti dove, evidentemente, il collegamento con il territorio rappresenta un fattore importante. Non mi dilungo su alcune

su cui la Commissione si è comunque impegnata, per andare invece ad una valutazione di carattere sintetico e complessivo. In questo quadro di criticità oggettive, oggettive, la fragilità del territorio, sia dal punto di vista morfologico che orografico, i porti di grandi e medie dimensioni e l'essere un territorio di confine sono elementi oggettivi di criticità. Vi è stata però una amplificazione di queste criticità per una mancanza di strategia complessiva, di inadeguata *governance* di sistema, di debolezza delle funzioni amministrative di verifica e di controllo. AIROLA *(M5S)*.

Come dicevo, le criticità presenti nel sistema ligure sono state purtroppo amplificate da una serie di fattori come la mancanza di una strategia complessiva, una debolezza delle funzioni amministrative di verifica

occorre agire in fretta, con atti concreti, sulla base delle linee strategiche che sono state tracciate, ma occorre anche la consapevolezza che nessuna scelta di carattere tecnico-organizzativo può essere di per sé risolutiva, senza l'ambizione e l'obiettivo di un nuovo patto che coinvolga istituzioni, imprenditoria e cittadini in un diverso approccio al tema dei rifiuti. Partecipazione, accesso alle informazioni, trasparenza, assunzione di responsabilità e innovazione sono i parametri su cui si misura la volontà di cambiare rotta di una classe dirigente. L'economia circolare, che ci impegna quasi a cancellare la nozione di rifiuto, ripensando radicalmente l'uso delle risorse, può essere, proprio per la Liguria, l'opportunità di un nuovo inizio nella gestione del ciclo dei rifiuti. Una Regione con un territorio dove si coniugano fragilità e bellezze e che ha l'accoglienza turistica nel suo DNA non può eludere una sfida che chiama direttamente in causa la qualità dell'ambiente. Una sfida che non può fare a meno dell'impegno, della concretezza e della serietà dei pubblici poteri in senso lato, ma anche della consapevolezza e della maturità dei cittadini e degli operatori economici*.

di intervenire perché non è tollerabile in quest'Aula che un collega si possa rivolgere a colleghi senatori con epiteti quali «assassini», «delinquenti», «criminali».

Senatore Airola, a questo punto lei deve lasciare l'Aula. Prego i senatori Questori di accompagnare il senatore Airola fuori dall'Aula, perché a questo punto ha superato ogni limite di comportamento*. (Applausi dal

nel sottosuolo che provocano quantità di rifiuti contaminati da amianto, anche in considerazione delle grandi opere in corso, non giustificano la grave situazione in cui versa la gestione dei rifiuti sul territorio regionale. Il ciclo rifiuti

non può venire davanti alla Presidenza a fare insulti in questi termini. La mia gestione è assolutamente equilibrata e paziente, anche troppo. Senatore Petrocelli, si accomodi.

PRESIDENTE. Io sto con il Regolamento e qua non è che si può insultare. C'è stata una tolleranza forse anche eccessiva, perché la dialettica esiste, l'insulto sistematico no.

di impiantistica. Non esistono termovalorizzatori, nonostante il fabbisogno di incenerimento sia di 235.000 tonnellate all'anno, e non esistono impianti di recupero, compostaggio e pretrattamento. La gestione dei rifiuti è invece fortemente dipendente da discariche, che oggi si trovano in esaurimento, e dal sistematico e dispendioso conferimento dei rifiuti fuori Regione sulla base di accordi interregionali. In Liguria vi sono dunque carenze persistenti, che nelle indagini condotte dalla Commissione risultano aggravate da un radicato sistema corruttivo, da forme di illegalità diffusa e anche da infiltrazioni criminali, che trovano terreno fertile proprio nella criticità del sistema. La mancanza per anni di una strategia complessiva sulla gestione dei rifiuti, che ovviamente ha delle responsabilità politiche ed amministrative locali ben precise, dove senza una programmazione per ambiti territoriali si sono delegati i Comuni, ha portato questo sistema inefficiente al limite del collasso. La situazione in Liguria è ancora più complicata, in primo luogo, dall'inadeguatezza alle normative di molti impianti di depurazione delle acque reflue urbane; in

dalle illiceità ipotizzate nella gestione della centrale elettrica Tirreno Power di Vado Ligure, non solo per l'inquinamento atmosferico prodotto dall'uso del carbone come combustibile, ma anche per per lo scarico delle acque e la gestione dei rifiuti. Infine, non mancano problemi nella gestione del SIN di Cogoleto-Stoppani, che impediscono gli interventi di bonifica ambientale. Una considerazione personale: la rilevazione dei problemi presenti in Liguria è frutto del grande lavoro svolto dal Corpo forestale dello Stato, un Corpo di polizia che, per decisione del Governo, dovrebbe essere in via di accorpamento nell'Arma dei carabinieri, ma che invece nei fatti è in via di disgregazione. Le ultime notizie che provengono dalla Conferenza unificata dello scorso 3 marzo - che sullo schema di decreto legislativo, quale delega della più ampia riforma della pubblica amministrazione, ha dato parere favorevole, ma subordinato alla possibilità per il personale di poter transitare nei Corpi forestali regionali e in quello delle Province autonome - è conferma di quanto la Lega Nord va sostenendo da un anno, cioè che siamo di fronte ad una vera e propria disgregazione del Corpo forestale, con gravi perdite di uomini, professionalità e competenze fondamentali per contrastare i danni all'ambiente e le frodi agroalimentari. Considerato che sono già intervenuto in sede di illustrazione delle relazioni del SIN di Porto Marghera e dei poli chimici del cosiddetto Quadrilatero, nei pochi minuti che mi restano esprimo alcune considerazioni sui rifiuti radioattivi, sui quali tornerò più ampiamente nella purtroppo unica dichiarazione di voto che sarà da me a questo tema completamente dedicata. Il tema della gestione dei rifiuti radioattivi e delle attività connesse rappresenta un esempio eclatante di alcuni dei problemi strutturali in cui versa il nostro Paese. I ritardi e i molteplici problemi evidenziati dalla Commissione riguardano: le attività di *decommissioning* degli impianti nucleari, l'individuazione del sito e la realizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi; la la capacità tecnico-gestionale della Società di gestione degli impianti nucleari (SOGIN), interamente pubblica e controllata dal MEF con funzioni di indirizzo del MISE; l'assenza del programma nazionale della gestione del combustibile nucleare, che secondo la direttiva Euratom doveva essere consegnato il 23 agosto 2015;

mettono in rilievo una situazione di paralisi delle procedure amministrative in corso, che espongono seriamente il nostro Paese a certe procedure europee La Commissione ha approfondito con adeguata cura la situazione, mettendo in risalto le carenze del sistema e, soprattutto, l'aumento dei costi determinati dall'allungamento dei programmi di *decommissioning*, che inevitabilmente ricadono sui clienti finali del sistema elettrico, essendo posti a carico della bolletta elettrica attraverso la componente tariffaria A2. da sottolineare come la riprogrammazione 2015 del *decommissioning,* rispetto a quella fatta nel 2010, porta ad allungare mediamente di ulteriori dieci anni il tempo necessario per lo smantellamento delle vecchie centrali e a far lievitare il costo previsto

Anche la Commissione ha espresso perplessità in ordine alla particolare severità che l'ISPRA ha assegnato al criterio di sismicità che, fatte salve parte di Lombardia e Piemonte, esclude sostanzialmente l'idoneità della quasi totalità del territorio nazionale per ospitare il Deposito nazionale. Si ritiene inoltre grave la scelta di non tenere conto degli aspetti idrologici ed idrogeologici del sito, che può dare luogo a una inaccettabile discrezionalità per la localizzazione del deposito. Mi avvio a concludere il mio intervento sul caso Cemerad di Statte, in Provincia di Taranto, che è un evidente esempio delle possibili conseguenze della cattiva gestione, a tutti i livelli, della situazione. In questo caso occorre un censimento su scala nazionale della presenza di depositi di sostanze radioattive, delle quantità immagazzinate, della loro localizzazione, dei processi attuati presso tali depositi, delle modalità di smaltimento finale utilizzate, delle garanzie tecniche e finanziarie in atto per impedire situazioni paragonabili a quelle che si sono venute a creare presso la Cemerad di Statte. Grazie all'intervento e all'azione della Commissione d'inchiesta, il Governo è intervenuto con cospicui Grazie anche per altre situazioni emergenti sul territorio nazionale, di valore ambientale, protezionistico e sociale non meno importanti, come ad esempio il caso Premoli di Rovello Porro. *(Applausi dal Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, in questo mio intervento commenterò i documenti nn. 9 e 11, ovvero le relazioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato di avanzamento dei lavori di bonifica nel sito di interesse nazionale di Venezia-Porto Marghera e sulla situazione delle bonifiche dei poli La bonifica del SIN di Venezia-Porto Marghera è sicuramente di particolare importanza e complessità, considerate soprattutto le specificità locali e le criticità che purtroppo non mancano. I lavori della Commissione hanno avuto obiettivi ambiziosi: da una parte, garantire una puntuale valutazione della situazione dei lavori di bonifica del sito, dall'altra ridefinire in modo ordinato e sistematico le procedure, nonché le soluzioni concrete emerse dai lavori di indagine. Gli approfondimenti emersi e contenuti nella relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, non solo sono preoccupanti, ma evidenziano come sia doveroso intervenire rapidamente sia a livello locale che nazionale. Mi preme ricordare, prima di tutto, che se fino alla metà degli anni Ottanta non c'è stato non c'è stato alcun controllo sulle diffusioni di sostanze provenienti dalle industrie di Porto Marghera, oggi vincoli nazionali ed internazionali inerenti sia al tipo che alle quantità degli scarichi impongono l'utilizzo di severe misure di controllo e riducono sensibilmente il potenziale inquinante di tutta la zona. La strategia di intervento per Porto Marghera ha le sue origini nell'accordo di programma siglato il 21 ottobre 1998 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel mese di febbraio del 1999. Tale strategia consisteva, fin dall'inizio, nell'isolamento mediante marginamento con palancole delle varie macroisole componenti il SIN, allo scopo di isolare le sorgenti di contaminazione ed evitare l'ulteriore apporto in laguna di acque di falda contaminate. Tuttavia, ad oggi, la bonifica, per la quale sono stati spesi finora circa 781 milioni di euro, corre il rischio di essere invalidata se i lavori non saranno completati secondo procedure ben precise. Ancora più sconcertante è il fatto che il mancato completamento di tali opere stia provocando il progressivo indebolimento anche dei tratti terminali delle strutture già realizzate e stia mettendo in serio dubbio la bontà complessiva degli interventi finora realizzati. Un altro aspetto da tenere in considerazione è la riqualificazione industriale che riguarda i 2.000 ettari di insediamenti produttivi, commerciali e terziari che fanno di Porto Marghera una delle più grandi zone industriali costiere d'Europa; difatti, l'inquinamento continua ad essere alimentato proprio dai tratti che non sono stati bonificati e, dunque, se non si farà in fretta - cosi come denuncia anche il presidente Bratti a capo della Commissione d'inchiesta di cui faccio parte - sarà una sciagura non solo finanziaria e economica, ma soprattutto ambientale perché l'inquinamento esistente si aggraverebbe. Gli enormi ritardi accumulati negli anni, a fronte di un rischio ambientale continuo ed elevato, sono stati approfonditi nella relazione sullo stato di inquinamento e dell'esposizione dell'area, dove si sono considerate soprattutto inadeguate le indagini fin qui condotte. Ne conviene che il finanziamento per interventi necessari di messa in sicurezza e per la bonifica delle aree non può essere più una scusante vista l'emergenza ambientale in atto. Passiamo ora alla relazione sul Quadrilatero, che ha coperto un maggior numero di SIN, ovvero le aree di Venezia-Porto Marghera, Ferrara, Mantova e Ravenna. In queste differenti aree la Commissione ha riscontrato situazioni ben diverse sia per il grado di inquinamento rilevato sia per la

Dal punto di vista tecnico, lo spettro di contaminanti riscontrati nei suoli e nelle acque sotterranee si presenta molto vario, posto che in molti casi è stata rilevata la presenza di diverse famiglie di contaminanti. In particolare, nei suoli sono stati rinvenuti metalli pesanti (arsenico, cromo, mercurio, nichel) e idrocarburi policiclici aromatici (IPA); nelle acque di falda sono stati rinvenuti metalli pesanti, IPA e composti organo-clorurati. Si tratta di un inquinamento grave sia dei suoli che delle acque di falda. La genesi di tale inquinamento è sostanzialmente dovuta a tre fattori: l'avanzamento della linea di costa, che è stato ottenuto impiegando rifiuti di lavorazione derivanti dalla prima zona industriale, sicché vi è stato un inquinamento da terreni di riporto; le emissioni incontrollate di varie sostanze, principalmente cloroderivati, tra i quali il cloruro di vinile e il PCB; la ricaduta degli inquinanti immessi nell'atmosfera nei corso degli anni. Dal punto di vista degli interventi è doveroso sottolineare che le azioni volte alla bonifica delle contaminazioni devono essere pianificate in modo puntuale e, solo a seguito di una dettagliata e rappresentativa caratterizzazione, devono essere portate avanti con impegno costante e non discontinuo. Le complesse e talvolta non trasparenti ripartizioni finanziarie delle risorse sono assolutamente da evitare, pena, senza dubbio, il rischio di vanificare gli impegni e le opere già eseguiti, con conseguente sperpero di denaro pubblico. La Commissione ha rilevato che l'ufficio del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, nella veste di committente dei lavori per conto dello Stato, non ha mai esercitato, né esercita tuttora alcun effettivo controllo sia sul sistema di assegnazione, da parte del consorzio Venezia nuova, dei subappalti relativi alle bonifiche, sia sulla congruità dei corrispettivi corrisposti alle ditte subappaltatrici. La carenza di controlli ha consentito al consorzio Venezia nuova di assegnare gli appalti alle ditte consorziate in violazione della normativa sulle gare d'appalto, del codice sui contratti pubblici e delle direttive europee. Dalla relazione emergono chiaramente tutte queste problematiche, che vanno anche a toccare il tema dei collaudi per cui sono stati stanziati rilevanti fondi, ottenendo, di contro, risultati esigui molto opinabili. Passando al SIN di Ferrara, che corrisponde all'attuale Polo chimico di Ferrara, denominato Stabilimento multisocietario petrolchimico, questi occupa nel suo complesso un'area di oltre 250 ettari, nella quale la concentrazione di attività connesse all'industria chimica ha determinato nel tempo fenomeni di contaminazione delle matrici del terreno e delle acque sotterranee. In questo caso, la bonifica dell'area è partita sostanzialmente in regime di decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, e poi proseguita tra il 2012 e il 2013 con la ridefinizione di un'analisi di rischio. Negli anni successivi vi sono stati aggiornamenti e approfondimenti di alcune fasi, sino agli anni 2014 e 2015. In questo caso, ha avuto un ruolo importante la IFM Ferrara ScpA, una società consortile costituita nel 2001-2002 dalle società insediate nello stabilimento multisocietario al fine di gestire i servizi. La possibilità di interfacciarsi efficacemente con l'esterno grazie all'esistenza di un soggetto unico consortile quale la IFM Ferrara ha comportato la redazione di piani di emergenza e lo svolgimento di esercitazioni con il coinvolgimento della popolazione. Sono previsti, dunque, un Piano di emergenza esterna (PEE) e l'attivazione di un Centro operativo misto (COM) e di un Centro operativo comunale Le società coinsediate hanno gestito autonomamente l'*iter* di bonifica delle rispettive matrici dei terreni e della falda, mentre il progetto di bonifica della falda confinata è stato gestito sin dall'inizio in maniera congiunta mediante lo strumento del consorzio IFM Ferrara. Stando alle dichiarazioni riportate nella relazione, i lavori stanno procedendo con efficacia. È importante segnalare che l'ARPA Emilia-Romagna è intervenuta positivamente in tutte le fasi della procedura di bonifica, con sopralluoghi e prelievi di campioni per validare i risultati raccolti dalle aziende durante le indagini e gli interventi eseguiti. Per quanto riguarda il SIN di Ravenna, si segnala che lungo il canale Candiano, che si estende per circa 11 chilometri collegando la città al mare, negli ultimi sessanta anni vi è stato un fortissimo sviluppo delle attività industriali; in particolare, a partire dagli anni Cinquanta si è sviluppato uno dei poli petrolchimici più importanti d'Italia. Le aziende che hanno maggiormente segnato il territorio sono quelle insediatesi nell'area dell'ex ANIC (ora Stabilimento multisocietario Versalis) e l'ex raffineria Sarom. L'area industriale presenta, quindi, situazioni di contaminazione derivante da epoche di scelte produttive con bassa attenzione ambientale. La tendenza costante nelle Conferenze di servizi di fronte a proposte progettuali delle aziende, sulla base della sostanza contaminante, è stata quella di ricorrere il meno possibile allo smaltimento *ex situ* in discarica. Sono state sempre privilegiate le tecnologie - che si sono notevolmente notevolmente evolute nell'ultimo decennio - di bonifica *in situ*, quali il *landfarming*, laddove la contaminazione fosse magari di origine organica e, quindi, degradabile, aiutando la flora batterica naturale con ceppi batterici non cancerogeni, o comunque certificati di non patogenicità,

la società Switch era delegata alla gestione di plastica, cartone e rifiuti pericolosi (frammentati in una serie di commesse pubbliche onorate solo in teoria). La Switch, secondo i pm, pur di incassare il massimo delle provvigioni faceva risultare una quota di differenziata vicina al 40 per cento, mentre agli occhi degli investigatori non superava il 10

incapace e va commissariata nella sua totalità. Adesso possiamo dire che l'ultima parte della Regione - non mi interessa di che parte politica sia - è lì da otto mesi e non possiamo ancora accusarla, ma tutto il resto della classe politica ligure,

Genova SpA; viene liquidata con il Comune di Genova che ha un debito di 15 milioni con la Fiera. Eppure si liquida la Fiera per farla convergere, con un'alchimia, in un'altra società che è la Porto Antico SpA.

posizione. Il sistema Liguria è crollato, ed è ben chiaro chi comandava in Liguria, tra la banca, qualcuno del centrosinistra, qualcuno del centrodestra, e qualcun altro ancora. Oggi è in atto in Liguria una battaglia per chi va a riprendersi il potere nella nostra Regione. Ci sono vari schieramenti e oggi, ad esempio, c'è anche tutta la posizione di Carige, della banca principale del nostro territorio, la cui maggioranza è stata da poco acquistata da un grande imprenditore genovese. Proprio in questi giorni c'è un gruppo internazionale, un fondo che si chiama Apollo,

Quello che nascerà sarà una banca che probabilmente non sarà più legata al territorio. Così come, sul sistema dei rifiuti, abbiamo una società, l'AMIU, che con l'inceneritore a Scarpino avrebbe potuto fare utili e la e la stiamo distruggendo, secondo me scientemente, per farla convergere dentro IREN, che diventerà il nostro padrone. Purtroppo abbiamo una persona onesta e brava, come tutti dicono (che secondo me è il minimo sindacale per chi fa politica), che è il sindaco Doria, che non è un giocatore di poker e si è trovato davanti gente con il pelo lungo un metro che lo hanno buttato fuori da IREN e ci hanno fottuto una società. Adesso non abbiamo neanche più quella. Quindi, paghiamo carissimo le tasse della spazzatura, ci portano via la società, chiudiamo la Fiera di Genova senza un progetto, con 15 milioni di debiti che il Comune ha nei confronti della Fiera e anche con problemi per i dipendenti. Non sappiamo se faremo il Salone Nautico ed Euroflora, che portavano ricchezza alla nostra città. Paghiamo 900 euro per andare da Genova a Roma; non abbiamo più un treno che ci metta meno di cinque ore per andare a Roma e un'ora e mezzo, un'ora e quaranta minuti per andare a Milano. Da che cosa dipende questo? Dal fatto che siamo degli incapaci!

che oggi sono crollati. Perché il Comune di Sanremo è il comune con il maggior numero di dipendenti pubblici per numero di abitanti? Perché Perché arrivavano dai 20 ai 30 milioni all'anno dagli utili del Casinò e allora via con il clientelismo: assumiamone mille! Adesso non ci sono più gli utili e il Comune fallirà. Questa è la situazione di una Regione che non ha una soluzione, perché se erano incapaci i politici di ieri saranno ancora più incapaci i politici di oggi, perché non abbiamo una classe politica e una classe dirigente-imprenditoriale. Abbiamo solo bisogno di essere annessi: l'unico progetto che può salvare la Regione sul versante

Arrivano due milioni e mezzo di croceristi, vengono i pullman a prenderli per portarli all'*outlet* di Serravalle, invece che portarli nei nostri negozi! Ma siamo proprio dei deficienti!

dei comandanti dei Carabinieri, devono arrivare alla città cui sono assegnati e non conoscere nessuno. Non devono arrivare lì, messi su dagli amici degli amici, per difendere le rendite di posizione, per farsi riassegnare le banchine, magari per sessant'anni, a dei prezzi vergognosi, cui manca uno zero in confronto al resto d'Europa. Questa è la situazione che potrebbe risollevare la Liguria. Dobbiamo essere invasi. Sono tantissime le situazioni disastrose della nostra Regione, che ha il peggiore PIL di tutto il Centro-Nord d'Italia

Signor Presidente, il lavoro complesso e dettagliato cui è giunta la Commissione bicamerale, con le relazioni oggi presentate, va ad inquadrarsi in una prospettiva di coerenza operativa, rispetto a quanto già compiuto dall'analoga Commissione nella precedente legislatura. Si tratta di un lavoro di continuità, che è opportuno leggere come un quadro d'insieme su tematiche apparentemente differenti, ma alle quali siamo chiamati a dare una risposta unica ed univoca. Queste relazioni ci parlano di anni persi, di scarso coordinamento istituzionale, di sperpero di denaro pubblico, di mancanza di strategia e di visione e, purtroppo, ci parlano anche di malaffare. Il lavoro d'inchiesta, seppur articolato in diverse tematiche, ha un filo conduttore e cioè l'incapacità del nostro Paese, purtroppo, di fare i conti con l'evoluzione dei processi industriali e con la necessità di recuperare, da un punto di vista ambientale, territori e spazi ampi e fortemente antropizzati. La drammatica situazione delle politiche sui rifiuti in Liguria, la necessità di risorse per la bonifica e il riuso del cosiddetto Quadrilatero del Nord, gli sprechi, le sovrapposizione e la burocrazia pesante e frenante delle vicende legate a Porto Marghera, investigate approfonditamente e documentate dai colleghi commissari, sono una fotografia che dobbiamo tenere ben ferma in mente come monito per le nostre politiche attive: per questo voglio ringraziare i colleghi della Commissione. Pertanto siamo ancora più convinti che, anche per dare una risposta alla «mancanza di una strategia complessiva sulla gestione dei rifiuti nella regione Liguria» come dice testualmente la relazione, questo Paese aveva bisogno di una programmazione pianificata e strategica, come previsto dall'articolo 35 del decreto sblocca Italia. Per questo siamo ancora più convinti che, anche per dare una risposta alle assunzioni di responsabilità di chi per anni ha inquinato il cosiddetto Quadrilatero del Nord o Porto Marghera, sia stato necessario approvare la nuova disciplina penale sugli ecoreati. È inoltre opportuno che la riflessione che oggi fa questa Assemblea si concentri sul tema annoso dello smaltimento dei rifiuti radioattivi. un tema che non può ritenersi completamente affrontato con l'approvazione della relazione in esame, che è però una tappa fondamentale in un percorso di approfondimento e di confronto con gli attori istituzionali e para-istituzionali coinvolti. La questione della ancora mancata localizzazione del deposito nazionale per lo stoccaggio delle scorie, disseminate in vari depositi provvisori, è da sempre considerata come il problema prioritario su questo versante. Innanzitutto ritengo utile che anche in questo contesto e alla luce di quanto emerge dalla relazione della Commissione ci si possa ancora interrogare sulla giustezza di alcune scelte di politica energetica, come quella di rinunciare al nucleare, anche alla luce degli impegni - anche durissimi - che il nostro Paese si è assunto, sottoscrivendo, praticamente con tutti gli Stati del mondo, l'Accordo di Parigi verso un'economia sempre meno schiava di fonti energetiche fossili. Su questo però, purtroppo, non si può tornare indietro e oggi ci troviamo a riflettere sui tempi del *decommissioning*, sui costi, sugli impatti ambientali e sociali di una scelta, come quella del sito nazionale di stoccaggio, difficile e delicata, ma ineludibile e strategica. Infatti, come emerge chiaramente anche in questa relazione, si è pienamente consapevoli delle criticità che condizioneranno questa procedura, soprattutto in termini di pregiudizio sociale nei confronti della collocazione di una struttura di tale valore e grande - lo voglio evidenziare - opportunità. In secondo luogo, la delicatezza dell'attuazione di procedure di questo tipo deve necessariamente comportare un livello di sicurezza, di trasparenza operativa e di capacità gestionale ed organizzativa adeguati. Infatti, come è stato ampiamente evidenziato, la quantità di rifiuti da gestire è significativa. Parliamo di circa 40.000 metri cubi di materiale attualmente presente nei siti provvisori che, a causa di vincoli normativi ed operativi e dalle complesse procedure di trattamento, rappresentano uno dei punti più deboli dell'intera catena operativa. Appare chiaro che, al di là delle difficoltà di individuazione di un sito definitivo, ciò che condiziona ancora il dibattito ed alimenta i dubbi va ricercato nella lentezza negli attuali cicli di *decommissioning* degli impianti nucleari esistenti, della scarsità di risorse e soprattutto nella permanente assenza di chiarezza sul sistema di controllo e sull'autorità competente. L'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, di cui non è stata ancora avviata la piena operatività, non può più rimanere un'intenzione sulla carta. L'ISPRA, come emerso chiaramente dalle audizioni, sta svolgendo un ruolo non suo. Lo fa bene e con il massimo impegno, ma senza strutture adeguate e purtroppo senza risorse idonee. È prioritario in questa prospettiva definire la vicenda dell'Isin, procedendo alla ratifica della nomina del suo direttore e avviandone l'attività, e programmare un forte e rinnovato coinvolgimento e una rafforzata responsabilità dei due soggetti tecnici coinvolti quali Sogin e l'ISPRA. appare prioritario consentire il superamento dello stallo operativo che continua a condizionare la Sogin, soprattutto per quanto attiene ai limiti attuali della sua *governance*, che di fatto impongono al Governo una

soprattutto in termini di operatività in progetti dì respiro internazionale che possono anche comportare un valore aggiunto in termini di credibilità e fiducia nei confronti della capacità del nostro Paese. Un ulteriore aspetto che è stato affrontato in questa sede afferisce al ritardo della pubblicazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee ad ospitare il deposito nazionale, e su questo punto, ribadendo quanto sopra detto, condivido pienamente la preoccupazione espressa nella relazione della Commissione, anche in ragione, come è stato chiaramente evidenziato, dell'effetto deleterio che i continui rinvii possono determinare sull'immagine di credibilità e di trasparenza dell'intera iniziativa. Come è stato ampiamente detto in precedenza, l'Italia ha recepito nel 2014 la direttiva europea che istituisce un quadro per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, trascurare il ritardo maturato sul fronte dell'obbligo di trasmissione alla Commissione europea del Piano nazionale previsto dalla direttiva stessa, anche in ragione degli impegni italiani con il decreto legislativo n. 45 del 2014, con il quale addirittura si stabiliva l'approvazione del Piano entro il 31 dicembre 2014 anticipandone dunque i termini. Una mancanza che, in un momento difficile come questo per l'Europa ed il mondo sul piano della sicurezza, abbiamo il dovere di sanare senza continuare a tergiversare. Pertanto, in conclusione, ritengo che il lavoro svolto finora sia da considerare certamente lodevole poiché ingloba in maniera chiara tutti i limiti, le criticità e le falle di un sistema, di cui però oggi si comincia ad essere veramente consapevoli. Ritengo che la priorità sia dare la giusta rilevanza a questi temi e dare ottemperanza agli impegni contratti, non solo per dare credibilità al nostro Paese, ma anche per dare giusta attenzione ad istanze di sicurezza che per troppo tempo sono state subordinate ad altre priorità ed immolate sull'altare della superficialità amministrativa,

al continuo dilagare di farneticanti populismi e alle banalizzazioni ecologiste improvvisate e confuse come quelle cui abbiamo assistito questa mattina.

L'eredità in uno degli ambienti più belli e fragili del pianeta è pesantissima: oltre 3.200 ettari di terreno coinvolti; solo la metà è rientrata nel sito di interesse nazionale; 1.621 ettari inquinati da arsenico, cromo, mercurio, nickel, idrocarburi policiclici e aromatici, cloruro di vinile, policloruro bifenile. Come è possibile? Signor Presidente, i veleni emessi in atmosfera non spariscono: ricadono al suolo e si accumulano. Altri sono stati immessi direttamente nel suolo e nelle acque. Materiali inquinanti sono stati addirittura depositati lungo le rive, al punto che si è visto avanzare il limite di costa. Abbiamo 35 miliardi di euro di danni ambientali, ma la via delle bonifiche

Il rapporto «Sentieri» ha evidenziato l'aumento di alcune casistiche tumorali tra i cittadini residenti. Ora serve uno studio epidemiologico mirato sugli impatti subiti da lavoratori e dalle persone più esposte. È dovuto il ripristino dell'ambiente per le generazioni future e va pagato fino in fondo. Purtroppo a Marghera la legge sui reati ambientali, fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle, che finalmente istituisce il reato di omessa bonifica, arriva tardi: le società responsabili sono giunte ad una transazione, hanno pagato una cifra ed è lo Stato, ora, a dover provvedere. Ma hanno pagato 565 milioni sui 781 finora spesi; il resto viene dal Ministero dell'ambiente, cioè dalle tasse degli italiani, e per questo la spesa doveva essere oculata.

commissariato per lo scandalo MOSE, abbia assegnato subappalti senza gara, senza nemmeno regole prefissate. Nessuno ha controllato che le cifre fossero adeguate. Come venivano fatti questi subappalti? Ne sono derivati interventi in ordine sparso e incompleto, ognuno però con il suo collaudo inutile. Anzi, utile a chi lo faceva: decine di commissioni di valutatori, a volte in conflitto di interessi o premiati per questo fondamentale lavoro con un posto di dirigente al Ministero, come nel caso di Gaia Checcucci. Ci sono costati un milione e mezzo, senza dirci nulla sul risultato atteso. Nell'accordo di programma era previsto un collaudo finale; solo quello potrà dirci se il complesso integrato di interventi funziona. è ora come una spugna, imbevuto di veleno. Si è cercato di isolarlo realizzando una rete di drenaggi che convogli le acque inquinate alla depurazione. finché l'opera non è completa metalli pesanti, idrocarburi, diossine e altre sostanze tossiche e cancerogene continuano a filtrare in laguna. E la contaminazione ambientale e i rischi sanitari per la popolazione si aggravano. Cosa manca, dunque, a completare questo intervento? Il 5 per cento dei lavori, ma costano il 30 per cento dell'intera opera, perché i costi sono lievitati e nessuno ha controllato gli appalti. I soldi sono finiti e mancano le opere più complesse e delicate. Lo Stato ha patteggiato con i privati una cifra inferiore ai costi; poi ha sprecato anche quel poco. I privati sono al sicuro, però, perché una clausola mette in chiaro che i privati non possono più risultare responsabili se lo Stato non provvede. Marghera, però, mancano 250 milioni, e se non si porta a termine il lavoro si rischia addirittura di compromettere le opere già attuate. Il Governo non ha preteso a sufficienza dai privati, e i fondi li deve trovare il Presidente del Consiglio, che si è permesso di rubare 300 milioni agli italiani. Chiedete ad un cittadino se lo spreco è o no furto legalizzato. Il Governo ha sprecato 300 milioni di euro rifiutando di accorpare il *referendum* contro le trivellazioni petrolifere alle elezioni amministrative; un *referendum* sacrosanto contro un'attività che rende nulla all'Italia, che ha le tasse minerarie irrisorie, ma compromette salute, pesca, agricoltura, turismo, che sono le nostre vere miniere. Renzi aveva paura di perdere le amministrative se tanta più gente fosse andata a votare e se il *referendum* raggiunge il *quorum*, perde anche la faccia; per questo ha voluto due elezioni distinte. Per garantire gli interessi delle *lobby* inquinanti del petrolio ha sprecato i soldi per riparare a Venezia i danni di un'altra *lobby* inquinante. Ora 250 milioni per Venezia, per il ripristino della laguna, li deve trovare.

onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, la relazione territoriale sulla Regione Liguria approvata dalla Commissione bicamerale di inchiesta sul ciclo dei rifiuti è il risultato di un'indagine approfondita, frutto delle numerose audizioni di vari soggetti, sia pubblici sia privati, dei sopralluoghi sui siti oggetto di interesse nonché dell'analisi dei 113 documenti acquisiti da varie fonti. Vorrei ringraziare i relatori e tutti i commissari per il lavoro svolto, non solo

complessiva sulla gestione dei rifiuti, a una gestione frammentata dell'attività di raccolta dei rifiuti, molto spesso lasciata ai Comuni, e quindi più permeabili, in singoli contesti, di interessi poco trasparenti; una gestione basata principalmente sul conferimento in discarica, con *deficit* di impianti di pretrattamento nonché con livelli bassi e non soddisfacenti di raccolta differenziata, a una dotazione impiantistica insufficiente, come è stato riportato giustamente dalla relazione. Questo per quanto riguarda la gestione dei rifiuti urbani. Problematicità si registrano anche nella gestione dei rifiuti speciali, in particolare per la produzione e gestione dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, dei rifiuti contaminati da amianto e delle terre e rocce da scavo, considerato anche l'avanzamento di grandi opere. È carente anche la gestione degli impianti per la depurazione delle acque reflue, mentre per quanto riguarda la situazione dei porti liguri, gli elementi raccolti dalla Commissione hanno evidenziato le dimensioni, rilevanti e in crescita, del fenomeno del traffico transfrontaliero di rifiuti. Commissione ecomafie Bratti dice che non c'è dubbio che l'assenza, da sempre, di una strategia regionale e le mancate scelte impiantistiche hanno portato alla proliferazione di fenomeni di carattere criminogeno (non necessariamente di stampo mafioso) quali, per esempio, attività corruttive della pubblica amministrazione. L'approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche e della legge regionale che modifica le competenze in materia di governo del ciclo dei rifiuti, da parte della precedente giunta Burlando, era il primo passo importante per il superamento - in linea con gli indirizzi europei e nazionali - delle criticità evidenziate nella relazione. Sugli stessi provvedimenti la Commissione d'inchiesta aveva, tuttavia, colto delle carenze che sicuramente possono tradursi in correttivi. Quello che mi preoccupa è che il nuovo Governo regionale, per dare un segnale di discontinuità con l'attività della Giunta precedente, renda nulli gli importanti passi fatti fino ad ora, con il pericolo che in Regione perduri ulteriormente questo stato di emergenza. i senatori Compagnone e Morgoni - è una Regione altamente urbanizzata, con produzione *pro capite* di rifiuti più elevata rispetto alla media nazionale che, per la sua posizione geografica e conformazione morfologica, registra la presenza di grandi porti e di grandi poli industriali (per la raffinazione del petrolio, per la cantieristica navale, per la produzione di energia), nonché di importanti attività turistico-commerciali. Per questo motivo, ogni politica di gestione e programmazione del ciclo dei dei rifiuti e delle bonifiche deve essere adeguata e commisurata a queste caratteristiche. L'approvazione, da parte del Parlamento, di una risoluzione su questa relazione può essere il punto di partenza per far sì che Governo centrale, Regione e enti territoriali interessati convergano sulle azioni da intraprendere, per rendere al più presto efficaci le misure previste dal Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche. Solo in questo modo si potrà portare la Liguria fuori dallo stato di emergenza che l'ha contraddistinta in questi anni e che è il terreno su cui si radicano l'illegalità e le infiltrazioni criminali. Come previsto dal Piano regionale, la Liguria potrebbe diventare la Regione pilota dove sperimentare misure più cogenti per un reale sviluppo dell'economia circolare, un'economia non più basata sul consumo

all'altezza del compito che gli è stato dato. Credo inoltre che gli accordi interregionali, anziché interrompersi dopo la chiusura della fase emergenziale, possano essere rinnovati sotto altre forme. Si potrebbe sperimentare una pianificazione interregionale; ci sono importanti realtà, nelle vicine Torino e Parma, dove poter far confluire poter far confluire il poco materiale che non si riuscirà a riciclare, senza la necessità di creare ulteriori impianti. non ho risparmiato niente alla mia Regione, che è una bella Regione. Sul merito delle questioni non ho risparmiato nulla ed ho ravvisato la necessità di vedere, insieme ai colleghi della Commissione, quelli che erano i punti critici. Non ho parlato di casinò, di barche, di annessione, di fiere e di mercati, attenendomi al merito. che ha fatto il senatore Maurizio Rossi sulla Regione Liguria non mi trovano assolutamente d'accordo; anzi, io credo che facciano male alla Liguria, dette in questo modo e in quest'Aula. Nella

storiche ed architettoniche e buone amministrazioni, città che sono amministrate bene, senatore Rossi. Quindi eviterei di fare propaganda inutile in questo consesso

«In data 18 febbraio 2016 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico hanno trasmesso uno schema di Programma nazionale al Dipartimento per le politiche europee per il successivo inoltro alla Commissione europea. Lo scorso 18 marzo sono state, inoltre, avviate le procedure propedeutiche alla consultazione pubblica per la Valutazione ambientale strategica».

ci mette nella condizione di poter vivere questo processo con meno ansia, considerato che il Ministero ha ripreso per mano la situazione e intende procedere.

le relazioni oggetto di discussione ci danno un quadro generale non felice in cui versa il nostro territorio. Il tema ambientale, infatti, è ancora una questione aperta nel nostro Paese: riguarda ogni Regione del nostro territorio e tocca ognuno di noi, ma vede noi, in quanto rappresentati del popolo, impegnati in prima persona ad assumerci responsabilità per iniziare ad invertire la rotta, compiendo scelte che saranno fondamentali in tema ambientale e nello smaltimento dei rifiuti. Le relazioni, oggetto di discussione, della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati fanno emergere quanto ancora ci sia da fare per giungere a quella svolta decisiva. L'attenzione deve rimanere altissima e il nostro impegno deve essere assoluto su uno degli aspetti centrali, quello legato allo smaltimento dei rifiuti. Si tratta di un lavoro minuzioso che deve essere fatto in sinergia con l'Europa, affinché non si parli più di rifiuti, ma di risorse da utilizzare: alla cosiddetta economia circolare, unica prospettiva possibile per contrastare i cambiamenti climatici e il surriscaldamento globale. Ancora oggi l'Italia subisce le procedure d'infrazione da parte dell'Unione europea per il mancato rispetto della normativa comunitaria sulla gestione dei rifiuti e delle discariche. Le sanzioni che arrivano dall'Unione europea mettono in evidenza come il Governo, anche su questo tema così delicato, non abbia agito in modo soddisfacente. A pagare saranno sempre i cittadini per le mancate bonifiche delle discariche (sono circa 185 quelle abusive) e l'ammenda da corrispondere all'Unione europea si aggira su circa 80 milioni Cari colleghi, abbiamo sprecato tante possibilità e ci sono ancora troppe questioni aperte. L'attività illecita sulla gestione dei rifiuti che si è registrata in Liguria, ma anche in altre zone del Paese è un fatto pesantissimo per il nostro territorio. Il problema relativo a Porto Marghera, sito produttivo che rientra nel Quadrilatero della chimica, settore strategico per l'Italia e dal quale dipende il futuro dell'industria, è frutto delle carenze e delle lentezze della macchina burocratica statale. Il processo di bonifica, partito dal 1998, non hai mai visto la luce e non ha ancora portato a risultati soddisfacenti. Dobbiamo comprendere come il progresso della chimica e della ricerca tecnologica in Italia siano strettamente correlate all'attuazione delle bonifiche. È da lì che dobbiamo partire o ripartire. I buoni propositi non bastano più. Una sana politica ambientale dovrebbe prevedere una fiscalità ambientale adeguata che incentivi le imprese del settore a sostenere strategie aziendali che vadano verso un'economia sostenibile e che limiti i sistemi di produzione inquinanti a grande impatto ambientale. Anche in questo caso, l'Italia rimane sempre un passo indietro. Altro tema cruciale è quello relativo alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Siamo ancora lontani dal raggiungere quello sviluppo dei trattamenti di raccolta che l'Europa ci impone e che il nostro pianeta ci chiede, ci implora. In molte Regioni, oltretutto, pur avendo delle tasse altissime sui rifiuti, i cittadini non ricevono un servizio adeguato e pagano il conto di una mala-gestione dello smaltimento e della raccolta dei rifiuti. Le immagini di tante città del Bel Paese sommerse dai rifiuti possono ancora portare l'Italia a brutte figure internazionali. La cattiva gestione delle pratiche di raccolta dei rifiuti e del relativo smaltimento possono causare un vero e proprio rischio per la salute umana e la salvaguardia dei cittadini. Il Governo, nonostante le buone intenzioni, è ancora molto lontano dal mettere in atto un piano di bonifica dei territori a rischio. Dovremmo accelerare una serie di procedure burocratiche.

Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, la protezione contro gli effetti nocivi delle radiazioni ionizzanti è stata esercitata nel tempo da una pluralità di strutture, ma da diversi anni a questa parte dall'ISPRA. iniziative che nel 2009, attraverso l'istituzione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare (ASN), avrebbero dovuto interrompere in Italia la parabola di decadenza dei servizi nazionali di radioprotezione, in pieno oblio dopo il *referendum* successivo all'incidente di Chernobyl del 1986, sono decadute dopo l'incidente di Fukushima del marzo 2011. L'ISPRA, nel frattempo, ha continuato ad esercitare in *prorogatio* le competenze nella materia in una condizione di crescente precarietà. Con la direttiva Euratom del 2011 è stato istituito l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), cioè l'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione che, in piena indipendenza e autorevolezza, avrebbe dovuto in questo ambito subentrare ad ISPRA. Peccato che il percorso di costituzione dell'ISIN, iniziato nell'ottobre 2014

le Commissioni parlamentari abbiano espresso a maggioranza parere favorevole sulla nomina, questa non è stata ratificata dal Consiglio dei ministri, che pur lo aveva proposto, e dal Presidente della Repubblica. Quale che siano le ragioni ufficiali del congelamento della procedura non è stato dichiarato. Si conoscono solo indiscrezioni di stampa che non sono state confermate né smentite da numerose interrogazioni parlamentari, alle quali il Governo mai risponde. Di fatto l'Esecutivo, ad oltre un anno e mezzo dalla designazione, sembra paralizzato. Questo è gravissimo, tenuto conto che la funzione di tutela che l'ISIN dovrebbe garantire allo Stato e ai cittadini e l'urgenza per la sua operatività passano in subordine rispetto all'importanza dell'attribuzione della specifica nomina. Mi rivolgo al rappresentante del Governo per dire che è illusorio il fatto che l'esercizio di tale funzione in proroga da parte dell'ISPRA sia sufficiente a garantire in modo accettabile i diritti dei cittadini in materia di sicurezza Non dimentichiamoci anche il rischio di attentati terroristici! Voglio ricordare che proprio oggi e domani a Washington si tiene il *summit* mondiale sulla sicurezza nucleare. Il tema di interesse, che sarà particolarmente trattato, riguarda la necessità di contrastare l'insorgere di un potenziale terrorismo nucleare (contro gli impianti nucleari e i siti di stoccaggio delle scorie), anche alla luce dei recenti fatti di Bruxelles che hanno acceso i riflettori sul serio rischio che si corre. Oggi le funzioni dell'ISIN in stallo sono esercitate, inerzialmente, da un ISPRA che è sempre più in crisi, in una parabola di esaurimento delle risorse nazionali in tema di radioprotezione, come peraltro candidamente ha sostenuto lo stesso direttore dell'ISPRA nell'audizione del 30 luglio 2015 presso la Commissione parlamentare «Non può non essere evidenziato alla Commissione che il personale tecnico del dipartimento nucleare dell'Istituto ammonta oggi a circa 35 funzionari, il 40 per cento lasceranno il lavoro per raggiunti limiti di età entro i prossimi cinque-sette anni». È preoccupante il divario tra gli importanti impegni che l'ISPRA dovrebbe assumere, seppur in *prorogatio*, e le risorse presenti e le prospettive di un ulteriore assottigliamento e dissipazione delle competenze residuali. Un impatto della grave situazione potrebbe essere già presente nelle attività dell'ISPRA. Ad esempio, la sua guida tecnica n. 29, che contiene i criteri per la localizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, dimentica che avrebbe dovuto trattare anche la gestione dei rifiuti ad alta attività. Questa è una criticità che si aggiunge a quella dei criteri assunti, che ho denunciato nel mio intervento in discussione generale. Per uscire da un'enunciazione apparentemente astratta di criticità ed illustrare concretamente solo alcune delle situazioni sul tappeto seriamente compromesse dal perdurante stato di precarietà istituzionale del settore, si ricorda quanto segue: l'esigenza di seguire le procedure di localizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi; la sorveglianza e il regime di autorizzazione sullo smantellamento delle centrali nucleari italiane, che continua ad accumulare un ritardo pesantissimo; la la presenza sul territorio nazionale di sorgenti radioattive industriali e medicali in uso in Italia e del trasporto dei materiali radioattivi, compresi depositi di rifiuti radioattivi abbandonati o in attesa di decisione sul loro destino (tra cui anche i numerosi micro depositi che si sono formati a seguito di incidenti presso aziende del ciclo del recupero dei metalli); la presenza a pochi chilometri dai confini nazionali di centrali nucleari in esercizio, in grado di generare devastanti effetti radiologici anche a centinaia di chilometri di distanza ed effetti rilevabili sino a migliaia di chilometri, come dimostrato dagli incidenti di Chernobyl e Fukushima. Per esempio, la centrale slovena di Krško, anziana e collocata in zona ad elevata sismicità, ne è l'esempio più eclatante, essendo, tra l'altro, la centrale estera più vicina ad una grande città italiana (137 chilometri da Trieste). Per quanto sopra espresso, in ordine alle precarie capacità nazionali in tema di sicurezza nucleare del nostro Paese, anche contro eventuali minacce terroristiche e calamità naturali, riteniamo che il Governo debba uscire dall'immobilismo e spiegare quali sono i motivi che impediscono l'effettiva costituzione ed operatività dell'ISIN e quando questo avverrà; quali sono i programmi per riportare gli organici destinati alle attività di radioprotezione in carico allo Stato, palesemente sottodimensionati e minati dal mancato rinnovamento generazionale, ad un livello minimo di accettabilità, indipendentemente dalle strutture (siano oggi l'ISPRA e domani l'ISIN) deputate ad esercitare tali competenze; i motivi dello stallo della discutibile procedura per la localizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. Serve trasparenza, condizione essenziale per la credibilità degli attori e per la serena - ripeto, serena - accettazione delle scelte da parte dei cittadini italiani. Inoltre, l'Esecutivo deve prendere atto del problema Sogin e risolverlo, visto che la perdurante crisi dei propri vertici aziendali impatta sul profondo ritardo nello smantellamento delle centrali nucleari italiane e dunque sulla bolletta degli italiani. Renzi, dunque, non si limiti oggi e domani a fare passerella al *summit* mondiale sulla sicurezza nucleare; non continui a fare lo struzzo che mette la testa sotto la sabbia; garantisca la sicurezza nucleare del nostro Paese rimuovendo i troppi e perduranti problemi denunciati nella relazione.

Signor Presidente, signora Sottosegretario, onorevoli senatori, come già ho avuto modo di illustrare in sede di discussione generale, i documenti al nostro esame, al di là di ogni strumentalizzazione politica, sono meritevoli d'attenzione e di sincero apprezzamento per la loro precisione e concretezza. Dico questo perché nel corso degli interventi precedenti ho ascoltato tanti contributi, ognuno con una propria visione d'insieme, pur tuttavia consapevoli della preoccupante situazione ambientale connessa al ciclo dei rifiuti e sugli illeciti ambientali ad essi correlati. Mentre in discussione generale ho soffermato la mia attenzione sui siti di Porto Marghera e del Quadrilatero della chimica del Nord, ora vorrei approfondire la situazione ligure e quella dello smaltimento dei rifiuti radioattivi. Più nel dettaglio, da un'analisi del documento relativo alla gestione dei rifiuti in Regione Liguria, emerge in maniera preponderante la mancanza di una strategia complessiva sulla gestione dei rifiuti, il che si ripercuote su una serie di ulteriori criticità. La gestione è delegata quasi interamente ai singoli Comuni, quando invece sarebbe preferibile un sistema legato a territori più vasti, soprattutto in una Regione come la Liguria, che ha caratteristiche morfologiche particolari e una elevata urbanizzazione. Proprio la gestione affidata ai Comuni può comportare rischi di fenomeni corruttivi e di infiltrazioni mafiose. Non va sottovalutato, poi, che la Liguria è una delle regioni con il più alto costo *pro capite* per la gestione, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, tanto da far ipotizzare un possibile intervento della sezione dì controllo della Corte dei conti. Rimanendo in tema di illegalità, i porti liguri sono caratterizzati dal crescente fenomeno del traffico transfrontaliere dei rifiuti, ad opera di soggetti stranieri spesso supportati da intermediari italiani che, eludendo la normativa nazionale sul trasferimento all'estero dei rifiuti, dirottano verso Paesi asiatici o africani soprattutto materie plastiche, apparecchiature elettroniche e le batterie per auto, contando su leggi più permissive nei Paesi di destinazione, dove non sono previste adeguate tutele ambientali. ambientali. Questa filiera impropria della gestione dei rifiuti ha ripercussioni sul circuito economico nazionale, in quanto vengono perse grandi quantità di materie che potrebbero essere destinate al riciclo, in una visione di economia circolare. Desta allarme anche la presenza della 'ndrangheta che è riuscita ad infiltrarsi nel tessuto sociale ed economico ligure, entrando negli appalti e subappalti di servizi, quali quelli destinati allo smaltimento dei rifiuti, come risulta da alcune inchieste condotte negli ultimi anni dalla magistratura. Ragionando in termini numerici, alla Legione Carabinieri della Liguria tra il 2010 e il 2014 sono state denunciate 651 attività illegali connesse al ciclo dei rifiuti. E ancora, secondo quanto rilevato da Legambiente, la Liguria è la prima Regione del Nord Italia per illegalità all'interno del ciclo dei rifiuti, con il 6 per cento delle infrazioni commesse. Nella relazione della nostra Commissione si evidenzia come il traffico illegale dei rifiuti potrebbe essere più efficacemente contrastato mediante una maggiore interazione (e una integrazione dei sistemi informativi) delle forze di polizia tradizionali, dei corpi dell'Agenzia delle dogane e della Capitaneria di porto. Un altro problema molto serio legato alla gestione dei rifiuti in Liguria deriva dalle scelte impiantistiche: infatti, la relazione evidenzia come nel corso del tempo si sia solo ipotizzata la realizzazione di strutture tecnologicamente tecnologicamente avanzate straordinarie, che avrebbero dovuto risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti, ma che di fatto non hanno mai visto la luce, lasciando il territorio esposto a più livelli di illiceità. Pertanto, la questione deve essere affrontata con urgenza, in quanto la produzione dei rifiuti in Liguria è già di per sé molto alta, circa il 14 per cento in più rispetto alla media nazionale, anche per la presenza dei turisti soprattutto nei Comuni costieri. La gestione dei rifiuti risente di una complessiva arretratezza del sistema. Sul territorio mancano impianti di incenerimento e di termovalorizzazione, pertanto i rifiuti urbani vengono smaltiti principalmente nelle discariche, molte delle quali hanno raggiunto l'esaurimento e non sono più in grado di garantire l'autonomia gestionale all'interno del territorio ligure. Inoltre, sono dei tutto assenti le discariche per per rifiuti pericolosi. Molti soggetti auditi in Commissione hanno, più esplicitamente, parlato di «collasso annunciato» nella gestione del ciclo dei rifiuti. La Liguria, infatti, in questi anni non è riuscita a creare una strategia gestionale dei rifiuti che la rendesse autonoma e che le permettesse di avere una programmazione a lungo termine: negli anni, in base ad accordi interregionali, i rifiuti sono stati sistematicamente conferiti al di fuori della regione. Ma questo sistema deve essere velocemente modificato. Altri nodi da sciogliere sono quelli degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane (che in molti casi non risultano adeguati) e quello dei siti industriali inquinati (molti dei quali sono ancora in attesa di bonifica). Per il superamento delle numerose criticità sin qui segnalate, concordo con quanto esplicitato nella relazione, laddove si auspica auspica l'efficacia del nuovo piano di gestione dei rifiuti, che presenta tuttavia alcune carenze. È prioritario, infine, intervenire sulla prevenzione, in quanto la risposta sanzionatoria dell'autorità giudiziaria interessa fenomeni talvolta irreparabili di inquinamento e danno ambientale. Più complessa è, invece, la questione affrontata nel documento relativo allo smaltimento in Italia dei rifiuti radioattivi e alle attività connesse. Nello specifico, gli argomenti trattati sono il *decomissioning* degli impianti industriali, il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, il programma nazionale per la gestione del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, previsto dalla direttiva 2011/70/Euratom direttiva 2011/70/Euratom e il caso del deposito Cemerad di Statte in provincia di Taranto. Occorre specificare che in Italia lo smantellamento dei rifiuti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi esistenti è affidata alla Sogin, società per azioni a capitale interamente pubblico. Come evidenziato nelle pagine della relazione, purtroppo le operazioni di *decomissioning* sino ad oggi hanno proceduto molto lentamente, il che ha comportato negli anni un aumento delle previsioni di spesa. Un nodo molto importante che ancora non è stato sciolto è quello relativo al sito dove trasferire i rifiuti radioattivi già esistenti all'interno dei singoli impianti e quelli generati con il loro smantellamento, nel quale i materiali dovranno essere conservati in condizioni di massima sicurezza. Giova ricordare che l'Italia, secondo quanto disposto dalla direttiva già citata, avrebbe dovuto predisporre entro il 23 agosto 2015 un programma nazionale per la gestione del combustibile nucleare irraggiato e dei rifiuti radioattivi. Nonostante il decreto legislativo n. 45 del 2014 predisponesse l'attuazione alla predetta direttiva, ad oggi la situazione è ancora irrisolta. Questa situazione non solo comporterebbe una procedura di infrazione, ma rinvierebbe ancora una volta una soluzione definitiva alla delicata questione. La relazione, infine, affronta la situazione del deposito con rifiuti radioattivi dell'ex Cemerad di Statte a pochi chilometri da Taranto. La Commissione ha appurato che il deposito fatiscente e palesemente esposto a qualsiasi tipo di evento ha necessitato di un intervento urgente

che oggettivamente non era in grado di sostenere spese tanto gravose per un compito così delicato come lo smaltimento di rifiuti radioattivi di origine ospedaliera e industriale. è rilevabile che le indagini, le ispezioni, la raccolta dei dati, nonché le relative relazioni finali dimostrano le fragilità del territorio e le conseguenze imprevedibili qualora noi non fossimo tempestivi a mettere in atto soluzioni concrete. La messa in sicurezza e le eventuali successive bonifiche dei siti in oggetto, rappresentano quindi non solo un dovere verso i territori che già fin troppo hanno sopportato ma, al contempo, una sfida dal punto di vista ambientale e sociale. Per questo motivo, il voto favorevole del gruppo Gruppo Per le Autonomie-PSI-MAIE è un voto di responsabilità ed è giustificato sia nel merito che nel metodo. Mi sia consentito, infine, sottolineare come le presenti risoluzioni siano frutto soprattutto dell'attenzione e della precisione con cui ha lavorato tutta la Commissione di inchiesta:

Il lavoro della Commissione sul ciclo dei rifiuti - che ringrazio - è stato assolutamente prezioso ed ha messo in luce, ahimè,

di tutto l'insieme della gestione dei rifiuti radioattivi. Quindi, ciò sta a significare che siamo davvero in una situazione molto pesante e critica per quanto riguarda la sicurezza

ha fatto riscontro un aumento delle previsioni di spesa, che sono passate dai 4,35 miliardi di euro, stimati nel 2006, ai 6,7 miliardi di euro stimati nel 2011.

Come dicevo, il programma quadriennale predisposto dalla Sogin presenta un quadro peggiorativo rispetto ai programmi precedenti. Inoltre vorrei sottolineare le

ruolo di ispettorato alla sicurezza nucleare, abbiamo una situazione di *prorogatio* per quanto riguarda le competenze dell'Istituto con situazioni anche gravi dal punto di vista del personale e dei finanziamenti, che sono state ben evidenziate nella relazione e anche in alcuni interventi dei colleghi che mi hanno preceduto. Tutto ciò sta comportando una situazione molto seria, che ha messo in evidenza - questo è chiarissimo anche nella relazione e nella risoluzione - i gravi ritardi che abbiamo accumulato. Adesso il Governo ha riferito che

la proposta di Carta delle aree potenzialmente idonee. Su tale questione, che interessa

stessa. Il 20 luglio, l'ISPRA ha trasmesso ai Ministeri le proprie valutazioni sull'aggiornamento finale della Carta prodotto dalla Sogin, ma da allora non vi è stata praticamente più notizia. Faccio riferimento anche a dei *question time* e alle interrogazioni perché anche allora (e cito un'interrogazione recente

e, quindi, dell'informazione e della partecipazione degli enti territoriali e locali dei cittadini si dilata nel tempo. Noi condividiamo tutte le preoccupazioni e chiediamo, da questo punto di vista, un impegno fortissimo da parte del Governo. Vorrei ricordare che l'accesso all'informazione e la partecipazione sono i due elementi centrali dei processi decisionali in materia ambientale, come riconosciuto dalla Convenzione di Aarhus sul diritto di accesso alle informazioni. Per la storia del nostro Paese, Paese, per quanto accaduto sulle scelte sbagliate di qualche anno fa, a maggior ragione è fondamentale il processo di coinvolgimento delle Regioni e degli enti territoriali, la trasparenza, l'accesso alle informazioni e la partecipazione dei cittadini; invece la Carta è ancora secretata. Questo, per noi, è un grande elemento di preoccupazione, non soltanto per i cittadini ma per tutti quanti i livelli istituzionali. Perciò servono, a questo punto, impegni seri da parte del Governo, per le questioni

per scelte che siano improntate alla competenza e all'autorevolezza per quanto riguarda il futuro dell'ISIN. Da questo punto di vista, vi sono riferimenti nelle premesse, nell'impegno e nella risoluzione. Noi dunque esprimiamo, come

che è fondamentale per noi la richiesta - che avanziamo da anni - di esclusione definitiva dai saldi contabilizzati, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, delle risorse destinate dagli enti locali

Su Porto Marghera la relazione ha evidenziato quali sono stati gli elementi (non solo critici, ma anche di più) verificatisi in tutti questi anni

esprimiamo la nostra soddisfazione per il dibattito che oggi si sta svolgendo, perché non è sempre scontato che relazioni su temi così rilevanti da parte delle Commissioni d'inchiesta siano, poi, discusse in maniera così seria e approfondita dall'Assemblea. Nella fattispecie, il dibattito odierno consente una discussione ampia e una maggiore trasparenza rispetto a situazioni di per sé problematiche, gravi e complesse, che insistono, peraltro, su tutto il territorio nazionale. L'obiettivo dell'Assemblea è sicuramente quello di cercare di porre, ancora di più, i riflettori su tali problematiche, per evitare che cadano nell'oblio e nelle lungaggini burocratiche. Pertanto, auspichiamo un'approvazione all'unanimità delle proposte di risoluzione, perché è di tutta evidenza che la tutela dell'ambiente non deve e non può conoscere divisioni politiche, ma unicamente la volontà comune di superare le criticità rilevate. In sintesi, parlerò solo di alcuni aspetti, perché evidentemente condivido pienamente l'intervento testé fatto, in discussione generale, dal collega senatore Di Biagio.

si corre il rischio che anche il lavoro fatto si ammalori e che quei marginamenti realizzati non tengano più e, di fatto, non servano a nulla. Di conseguenza, vi è il rischio che lo scarso funzionamento delle strutture fin qui realizzate possa contribuire non a ridurre, ma addirittura ad aumentare il livello di inquinamento presente. La situazione attuale è, dunque, di una delicatezza estrema e chiama tutti ad un senso di responsabilità, al di là delle colpe di chi non ha realizzato in maniera adeguata un'opera o un'altra. Il rischio, appunto, è che continui l'inquinamento e che si possa riaprire un contenzioso tra lo Stato e le imprese che hanno pagato, attraverso transazioni, il corrispettivo per addivenire all'emergenza delle bonifiche e questo rischio - lo sottolineo - è molto forte e fondato. Inoltre, qualsiasi opera di reindustrializzazione venisse mai realizzata in quell'area (e ci sono tanti interessi manifestati, perché quella è un'area strategica, non solo per l'allocazione, ma anche per la sua naturale infrastrutturazione e per il naturale punto di approdo tra terra e non può non considerare la bonifica e la messa in sicurezza quale necessaria premessa. Quindi, bonifica e messa in sicurezza rappresentano la premessa del rilancio di un'attività produttiva e vanno assolutamente considerate di pari passo. Per quanto riguarda la bonifica dei poli chimici, il cosiddetto quadrilatero del Nord, che comprende, oltre a Porto Marghera, i siti di Mantova, Ravenna e Ferrara, dobbiamo ricordare che questo rappresenta il sito d'elezione della chimica italiana del Novecento: di quella chimica che ha dato risultati straordinari nel nostro Paese. La maggiore criticità riscontrate nei vari siti di interesse nazionale è la presenza di numerosi procedimenti amministrativi. A volte le imprese adducono questa complessità come una impossibilità per poter procedere a bonificare o mettere in sicurezza; a volte il pubblico scarica le responsabilità dicendo che non ha i mezzi per poter fare controlli Quindi, si tratta di normative che sicuramente necessitano ancora di essere perfezionate, anche se nel collegato ambientale, con l'approvazione di un nuovo schema delle transazioni finalizzate al ripristino ambientale, si è cercato di perseguire la logica delle semplificazioni. Parimenti importante è stata l'introduzione nel codice penale del reato di omessa bonifica, che sicuramente sarà una leva importante in mano alla magistratura per far rispettare i procedimenti in atto di messa in sicurezza e bonifica. Non ultimo, anche l'approvazione definitiva da parte del Senato della legge sul riordino delle agenzie ambientali potrebbe favorire questo processo di semplificazione. Al di là delle peculiarità dei singoli siti, che vanno assolutamente considerate, emerge di fatto che le bonifiche sono fondamentali se si pensa che in questi siti, oggi tutti attivi, la chimica del nostro Paese possa avere ancora un futuro, e non soltanto la chimica tradizionale. Versalis ha un centro di ricerca importante: un centro di eccellenza è a Ravenna e a Ferrara vi è il centro studi più importante per la produzione di poliolefine in Europa; a Mantova vi è un altro pezzo importante della ricerca di Versalis e vi sono anche siti che stanno guardando con un certo interesse a possibili investimenti sulla cosiddetta chimica verde. Ricordiamo che tanti brevetti innovativi, legati al cosiddetto *bio-based*, cioè alla cosiddetta chimica verde, sono in realtà frutto della ricerca italiana. Speriamo tutti che il nostro dibattito serva anche da stimolo per affrontare una discussione in tal senso per far sì che il Governo scelga, nella maniera giusta e opportuna, la via per rilanciare questa importantissima branca dell'economia nazionale. Per la prosecuzione delle attività di bonifica si richiede, dunque, non solo la destinazione di risorse economiche ma anche un ruolo attivo della parte pubblica, e mi riferisco in primo luogo del Ministero dell'ambiente, del Ministero dell'ambiente, che evidentemente deve riappropriarsi delle proprie competenze, delle proprie specificità e del proprio ruolo nel perseguire non una logica meramente procedurale ma una logica di risultato, dimostrando la capacità di coniugare, nell'interlocuzione con gli enti territoriali e i soggetti privati, elevate competenze tecniche e giuridiche e soprattutto capacità di visione strategica condivisa. Sulla questione del ciclo dei rifiuti in Liguria posso rifarmi agli interventi dei colleghi, ancora una volta del collega Di Biagio, ma sottoscrivo anche buona parte dell'intervento del collega Caleo.

Liguria, fa sì che quella rappresenti di per sé un'emergenza nazionale, magari misconosciuta. Si parla spesso di Meridione d'Italia, si parla spesso di Napoli, di Campania e di Sicilia, ma quella della Liguria è sicuramente una tematica sulla quale dobbiamo lavorare con maggiore incisività. Per non parlare, poi, delle grandi aree portuali che insistono in quella Regione, che costituiscono di per sé un punto di smistamento transfrontaliero di rifiuti non sempre leciti, anzi molto spesso addirittura illeciti, anche quando la regia di traffici illeciti si trova in altre parti del territorio nazionale: regia che evidentemente sceglie come porti di elezione probabilmente i porti della Liguria. Bisogna anche accennare alla questione della demolizione della Costa Concordia: un'attività di demolizione che, in considerazione della sua elevata complessità, nonché dei possibili, potenziali impatti ambientali, è stata preventivamente sottoposta all'Autorizzazione integrata ambientale e fatta oggetto di monitoraggio e controllo da parte del personale della Capitaneria di porto di Genova. Il caso Concordia è un caso eclatante, ma non deve essere considerato un caso unico. Ogni anno venti navi di grandi dimensioni vengono abbandonate nei porti italiani, anche perché sono iscritte nei registri navali farlocchi di Paesi compiacenti, con l'impossibilità di risalire alla titolarità di quelle imbarcazioni. A queste si aggiungono altri

ben 42.000 tonnellate di vetroresina. È un fenomeno rilevante, per il quale è ormai necessario provvedere con una specifica procedura di smantellamento dei relitti, salvaguardando l'ambiente e la sicurezza della navigazione. Per concludere, signor Presidente, ci sono da sottolineare gli aspetti più rilevanti in tema di gestione dei rifiuti radioattivi in Italia. La criticità fondamentale risiede nella perdurante mancanza di un deposito nazionale ove collocare i rifiuti, oggi distribuiti in numerosi siti sparsi sul territorio nazionale, in massima parte addirittura nelle aree dove gli stessi rifiuti sono stati prodotti. Di certo non giova alla fattibilità dell'opera il prolungarsi dei tempi di attesa per la pubblicazione della proposta della Carta delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Deposito nazionale, soprattutto per l'effetto negativo che i successivi, ripetuti rinvii possono produrre sull'immagine di trasparenza del procedimento, condizione indispensabile, insieme alla credibilità degli attori, affinché l'opera possa essere realizzata in un clima di sufficiente accettazione da parte delle amministrazioni locali.

all'esame quattro relazioni molto diverse tra loro che, nell'insieme, danno però tutte un quadro molto sconfortante della gestione e della sicurezza dei nostri territori. L'Italia che ne viene fuori è un'Italia approssimata e troppo spesso disonesta: non investe nella riqualificazione dei propri territori, a danno dell'ambiente e della salute, sì, ma anche della riconversione dei territori stessi e quindi della nuova economia. un Paese che non rispetta gli impegni di spesa e le scadenze e che non appare né affidabile, né efficiente. La prima relazione è relativa all'annosa questione della gestione dei rifiuti radioattivi, che già abbiamo trattato in 13ª Commissione, insieme alla 10ª legislatura precedente la Commissione bicamerale la definì una situazione sconfortante e non molto è cambiato. Le criticità principali che si leggono nella relazione sono la mancanza del deposito nazionale, che chiaramente, a catena, fa emergere tanti altri problemi e non consente una stabile messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, che sono ancora nei luoghi dove sono stati prodotti senza essere messi in sicurezza secondo gli *standard* attuali. Tra l'altro - e non è cosa da poco - questi potrebbero diventare obiettivi strategici per degli attentati terroristici, sicuramente catastrofici. La relazione rende incerta la prospettiva per le operazioni di *decommissioning* e quindi per rilasciare gli attuali siti nucleari liberi da ogni vincolo di natura radiologica, affinché siano riconvertiti la questione dei rifiuti prodotti nell'industria, nella ricerca e nella sanità, che vengono ad oggi raccolti in modo molto precario in depositi temporanei. inoltre non dà una destinazione per i rifiuti radioattivi prodotti con le operazioni di trattamento del combustibile irraggiato, che vengono condotte in Francia e in Gran Bretagna. l'acquisizione di questi prodotti, proprio perché non c'è il deposito e quindi non c'è sicurezza che questi rifiuti potranno essere riaccolti da noi entro il 2025, come previsto dall'accordo da noi sottoscritto.

quasi tutte interne alla Sogin stessa, che invece cerca di sminuire le proprie responsabilità. Un'altra importante criticità risiede nelle funzioni di controllo, che dal 1994 erano in capo all'ISPRA, che aveva le competenze adatte; dal 2009 si prevedeva di spostarle a un altro ente, ma tale spostamento non è mai avvenuto. La situazione di precarietà inevitabile per il periodo transitorio

molto arretrato, quindi ci saranno altri ritardi e dunque tagli, ma ritardi e tagli significano aumento di spesa, che è già di diversi miliardi. Tutte queste spese, però, sono a carico dell'utente elettrico tramite la classica, vecchia bolletta bolletta elettrica attraverso la componente tariffaria A2 e senza un tetto massimo predefinito, quindi questa cifra può aumentare senza che alcuno metta un limite. A peggiorare la situazione e la percezione negativa e sconfortante di questa situazione è il fatto che il presidente Zollino e l'amministratore delegato Casale, sentiti

anche a mezzo di una suggestiva campagna pubblicitaria, a settembre 2015, ma che continua a essere assolutamente riservata. Ci preoccupa molto che ciò non sia una premessa a una soluzione imposta e non condivisa, come era stato annunciato; una soluzione che quindi non potremo assolutamente mai accettare.

ma con parecchi mesi di ritardo, visto che era atteso per il 23 agosto. Naturalmente tutto quanto esposto non può non destare preoccupazione in merito ai delicatissimi compiti della Sogin

di alcune problematiche specifiche sui siti che sono veramente allarmanti. Non sono tuttavia più rassicuranti le conclusioni che ci offrono le relazioni sul cosiddetto quadrilatero della chimica e nello specifico su Porto Marghera. Il tema delle bonifiche è imbarazzante, perché riguarda più di mezzo secolo di inquinamento impunito e profondo dei siti, che ancora in questo momento sono inutilizzati e abbandonati e in cui l'inquinamento è attivo è attivo e devasta le falde acquifere superficiali e profonde, nonché la qualità dell'aria, perché l'inquinamento è un'azione attiva,

assoluto, sempre sottomesso al concetto del profitto e dell'imprenditoria, che invece è limitato costituzionalmente alla funzione sociale e all'interesse generale. Ma questo purtroppo accade

si è voluto credere che le bonifiche non avvenissero per la complessità dei controlli e si è tagliato sui medesimi. Nel decreto competitività, per esempio, nel giugno 2014 si è introdotta l'autocertificazione dello stato di inquinamento del soggetto interessato e il silenzio assenso sui piani di caratterizzazione di privati, senza contraddittorio dell'ente di controllo. Tutto ciò avviene nel Paese

per definirlo. La laguna e le acque intorno al petrolchimico sono devastate dai veleni. Il primo accordo di programma è di diciotto anni fa, però la laguna di Venezia

incompiuta e dei contenimenti non realizzati a regola d'arte. Forse andranno perduti 781 milioni, di cui 500 sono transazioni

Importante è vedere come siano stati assegnati ad assessori e dirigenti apicali della Regione Veneto, a *ex* capi gabinetto del Ministro dell'ambiente, a direttori generali del Ministero dell'ambiente, a figure apicali del magistrato delle acque di Venezia,

forse sono create allo specifico scopo di permettere illeciti. Emerge una mancanza di strategia complessiva di gestione dei rifiuti urbani e di quelli pericolosi. Ancora il 60 per cento va in discarica

Da allora questa Commissione è andata ad affiancare Commissioni bicamerali storiche come, ad esempio, la cosiddetta Commissione antimafia. La mafia esiste ancora e su di essa ancora si indaga. Anche la Commissione d'inchiesta sui rifiuti è costretta ad indagare e predisporre studi, analisi ed approfondimenti territoriali e tematici sulle tante forme di smaltimento illecito dei rifiuti. Le anomalie di comportamento e la violazione sistematica della legge e delle pratiche consentite sono alla base dell'esigenza di dare corpo ad ogni legislatura a questo organismo bicamerale, con la consapevolezza che le problematiche legate al ciclo dei rifiuti sembrano sempre più collegarsi ai problemi trattati anche nell'altra Commissione bicamerale, cui ho fatto cenno. Il problema rifiuti si intreccia ogni giorno di più con la criminalità organizzata, che vede nella gestione dello smaltimento una ricca occasione per fare profitti. Molte aziende che si occupano di smaltimento rifiuti sono risultate collegate alla criminalità, storicamente legata alle imprese che si occupano dei lavori di movimento di terra e cave realizzati con camion, pale meccaniche e ruspe, con centinaia di denunce registrate negli ultimi anni. Si è creato, quindi, un legame quasi automatico con la nuova tipologia di attività legata allo smaltimento dei rifiuti e tanti sono stati i casi di appalti truccati o pilotati pilotati finiti nel mirino della magistratura, tante le condanne e tanti i procedimenti penali in corso. La Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti si è occupata anche di questo, fornendo una fotografia recente e nitida del fenomeno. Riconosciamo volentieri che enorme e prezioso è stato l'impegno in audizioni, sopralluoghi e acquisizioni di materiale, utilissimo ad approfondire le tematiche trattate. Ora è necessario fare tesoro di tutta l'attività svolta, conferendo concretezza ed operatività al lavoro compiuto. Rispetto all'estesa indagine svolta, è possibile, nella brevità di una dichiarazione di voto, accennare solo a qualche punto. I quattro documenti al nostro esame ci consegnano tematiche in parte differenti. Vi sono infatti il documento che riguarda la gestioni dei rifiuti radioattivi due documenti che trattano le bonifiche di siti industriali, tra cui i poli chimici, partendo da un documento approvato dalla Commissione nel dicembre scorso, che riguarda Venezia e Porto Marghera, per arrivare a ricomprendere il cosiddetto quadrilatero del Nord, che include Mantova, Ferrara e Ravenna nel documento approvato appena un mese fa.

giustizia e, poi, del Procuratore nazionale antimafia, del Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e di decine di rappresentanti della magistratura e delle Forze dell'ordine ai massimi livelli di responsabilità territoriale. A nostro avviso, pur valutando positivamente le importanti relazioni consegnate al dibattito odierno dell'Assemblea del Senato, sarebbe necessario trarre da esse articolate conclusioni operative che possano essere valide a livello nazionale e che divengano la base per la pianificazione di un intervento strutturato di settore, a partire dalla relazione sulla gestione dei rifiuti radioattivi in Italia, che - va ricordato - non sono solo i materiali radioattivi usati negli impianti nucleari ormai dismessi, ma anche una parte dei rifiuti ospedalieri, dell'industria e dei laboratori di ricerca. La relazione fotografa lo stato dei fatti per la gestione del Deposito nazionale, problema che si trascina da anni senza soluzione. Non dimentichiamo che una componente della tariffa della bolletta elettrica (per la precisione,

quest'ultima in attesa di trasferire funzioni e relativo personale a ISIN, superando la recente pessima figura del Governo, al fine di garantire l'efficace espletamento della richiesta a funzione di controllo. Probabilmente la soluzione potrebbe essere quella di legare la realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi a un importante centro di ricerca in materia. Se questo è lo scopo dell'ipotizzato parco tecnologico, guardiamo con favore a questa proposta. Tale soluzione potrebbe forse contribuire a superare i tanti ostacoli frapposti da parte delle comunità locali all'individuazione e realizzazione del sito. Se si crea un centro di eccellenza nella ricerca nucleare e si consegna una garanzia di assoluta sicurezza e di trasparenza alle comunità sulla gestione dei rifiuti radioattivi, sul piatto della bilancia potrebbero essere più i vantaggi rispetto agli svantaggi per la realizzazione del sito. Senza considerare che è stato calcolato che ulteriori ritardi nella realizzazione del deposito potrebbero portare comunque a un costo di circa un miliardo in un decennio in penali da pagare a carico dell'Italia. Quindi su questo tema servirebbe una maggiore capacità decisionale da parte del Governo, che porti a una soluzione veloce e trasparente non più procrastinabile. Nell'approccio al settore dei rifiuti radioattivi ci si trova insomma di fronte a un'ordinaria storia di ritardi accumulati (gli ultimi a partire dal decreto‑legislativo con una serie di danni a cascata causati dall'assenza di decisioni operative, *in primis* l'insostenibile ritardo nella formulazione della proposta contenuta nella Carta delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del deposito nazionale. Costituiscono un'importante analisi anche le due relazioni sui lavori di bonifica dei poli chimici del cosiddetto Quadrilatero del Nord. Condividiamo l'esigenza di coniugare la necessità della bonifica

che sono state individuate quali barriere alle prospettive di reindustrializzazione. Andrebbe realizzato un miglior utilizzo dei fondi pubblici a disposizione per le bonifiche, attraverso l'esercizio di un effettivo controllo tecnico-amministrativo sugli interventi da completare a partire, ad esempio, dai marginamenti delle macroisole di Porto Marghera, attraverso un maggior coinvolgimento del ruolo e delle risorse dei privati e uno snellimento delle procedure di bonifica e per il riutilizzo del sito per scopi successivi, a partire dall'esigenza amministrativa di organizzare i numerosi enti interessati attraverso un forte coordinamento, dotato di competenze e conoscenze adeguate alla complessità delle materie da affrontare. Per quanto riguarda la relazione sulla Liguria, siamo in presenza di una ricognizione ampia delle situazioni in essere e delle diverse problematiche rilevate dalla Commissione

sono particolarmente difficili da tenere sotto controllo. Tra l'altro, incide la stagionalità dei rifiuti solidi urbani in una Regione a vocazione turistica che vede ampliata la popolazione presente soprattutto nei mesi che vedono la maggiore affluenza dei visitatori.

il nuovo sistema di accesso alle banche dati ambientali del sistema informativo regionale, rendendo quindi più chiara la situazione regionale, archiviando le informazioni derivanti dai controlli e dai monitoraggi ambientali. Relativamente alla relazione territoriale sulla Regione Liguria, reputo che uno dei punti di grande merito della Commissione sia l'aver portato nell'Aula del Senato, senza ammorbidimento alcuno, una questione di particolare rilevanza nella gestione delle emissioni e dei rifiuti che attiene alla produzione di energia nella centrale termoelettrica Tirreno Power di Vado Ligure, caratterizzata da una sistematica azione dolosa nei confronti del territorio. Lo dico perché questo vero disastro (in cui avrebbero perso la vita, a causa di condotte illecite di gestori e di funzionari pubblici, non meno di quattrocento persone, e sarebbero state trattate in modo illecito più di 27.000 tonnellate di rifiuti) deve essere analizzato, nel rispetto dell'azione in corso da parte della magistratura, sino in fondo, in modo da permettere l'individuazione di procedure e modelli gestionali adeguati tecnicamente ed amministrativamente alla gestione di siti industriali complessi, superando commistioni politica-affari-istituzioni che hanno segnato pesantemente la Provincia di Savona per lunghi anni. L'argomento non può essere compresso in una breve discussione e richiede certamente un approfondito esame, di cui lo specifico capitolo della relazione può costituire la base di partenza. Concludo, signor Presidente, valutando positivamente le relazioni della Commissione bicamerale e invitando il Governo a raccogliere le pur succinte indicazioni che abbiamo segnalato in questa nostra dichiarazione di voto, con l'ulteriore sollecitazione a procedere con azioni concrete, utili a garantire la sicurezza dei cittadini e delle imprese, nel settore del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti in modo di evitare ulteriori esborsi a causa di dannosissime procedure di infrazione. Il Gruppo di Forza Italia voterà a favore delle quattro risoluzioni, con l'auspicio finale che l'impegno richiesto al Governo non resti lettera morta e porti rapidamente verso soluzioni adeguate.

potuto e dovuto permettere ciò che è accaduto in quest'Aula, con gli epiteti e gli insulti che abbiamo ascoltato. Credo infatti che chi ha affrontato seriamente questi temi

abbiamo visto un'Italia che vuole risollevare lo spirito, risolvere i problemi e mettere al centro la legalità, vuole fare della trasparenza e della certezza del diritto la

relativi ai marginamenti della laguna di Venezia. Ci siamo resi conto, leggendo le carte, che tutte quelle figure erano state in larga parte compensate di un ruolo duplice di controllato e controllore, con ciò diluendo le le penalizzazioni che avrebbero dovuto essere poste a capo dei responsabili. Questa è una Commissione che, laddove

che questo Parlamento ha nelle Commissioni d'inchiesta uno strumento fondamentale, non solo per permettere che le leggi che in questo Parlamento, in questo Senato, vengono approvate, divengano operatività e azione positiva per i territori, ma anche per permettere di rendere, come stiamo facendo oggi, un *report* ispettivo delle inchieste che siamo andati a

C'è un'Italia che non ha funzionato, in Liguria, nel Lazio, in Toscana e in molte altre parti della penisola, ma c'è anche un'Italia che funziona. quello che è avvenuto all'interno dei SIN di Ferrara e Ravenna ci permette di dire che, dove c'è una *governance* pubblica in grado di prendere per mano il complesso sistema delle bonifiche insieme con le imprese private che vogliono attuare quelle bonifiche per reindustrializzare aree altrimenti malate, i SIN funzionano e possono procedere.

ci permette di attivare un settore industriale tecnologicamente molto avanzato, nel quale l'Italia ha potenzialità per consolidare competenze e eccellenze pienamente e massicciamente spendibili nel panorama industriale internazionale. Sono già 10 gli impianti che si sono spenti nel resto d'Europa. Se facessimo valere il nostro *know how* e le nostre potenzialità,

e precisando che il lavoro che vorrei che la politica svolgesse non è solo quello dell'accusa in quanto tale, che serve sì, ma serve a poco, ma anche quello di accendere una candela quando c'è il buio e cioè di permettere che si proceda

l'idea di istituzioni malate, che non funzionano, che litigano, che si contrastano con parole ingiuriose quando invece ciò che abbiamo fatto stamane

Signor Presidente, intervengo in dissenso sul solo documento n. 7, che riguarda la relazione sulla gestione dei rifiuti radioattivi in Italia. l'impegno e anche le osservazioni dei miei colleghi del Movimento 5 Stelle, che hanno svolto un ottimo lavoro in Commissione, e anche i rilievi giustamente critici della Commissione tutta. le richieste che si fanno in questo documento siano troppo deboli, limitandosi ad espressioni di preoccupazioni o di auspici. Cito brevemente due punti in particolare che mi hanno lasciato perplesso. Uno è l'ampia disquisizione che la Commissione ha fatto sul criterio per cui l'ISPRA, nel giugno 2014, basandosi sui dati dell'Istituto di geofisica e vulcanologia, ha praticamente indicato indicato l'opportunità di escludere, con il solo criterio della sismicità elevata, quasi tutta l'Italia dall'individuazione del sito per lo stoccaggio delle scorie nucleari.

di geofisica e vulcanologia, ad esempio di tipo sociopolitico o socioeconomico. Pensiamo, alla luce dei recenti attentati in Belgio, all'ipotesi di un trasporto via mare di scorie nucleari: credo che vi sarebbero grossi problemi, anche dal punto di vista di possibili rischi di possibili rischi terroristici. Per non parlare dell'ipotesi assurda di situare uno stoccaggio di rifiuti nucleari in Regioni in cui si svolgono esercitazioni militari, dove ogni tanto qualche missile sfugge al controllo (mi riferisco alla mia Regione, la Sardegna). Altre considerazioni sono state ignorate dalla Commissione, come quelle socioeconomiche, concernenti l'incompatibilità di determinate attività economiche - penso a quelle turistiche - con la presenza di un sito di rifiuti radioattivi. Ma la cosa che più mi ha fatto propendere per il voto contrario è stata la mancata richiesta di una correzione del decreto legislativo n. 31 del 2010, che prevede, sì, come privilegiata una procedura condivisa di individuazione del sito, ma non esclude, come invece avrebbe dovuto fare, l'ipotesi di ricorrere ad una procedura impositiva in caso di fallimento di un'intesa. In un territorio in cui si deve praticamente mettere un vincolo eterno (perché stoccare scorie nucleari significa avere in quel territorio un vincolo eterno) non si può assolutamente ipotizzare una procedura impositiva, a costo di pagare tutti noi, tutto il resto d'Italia. In quel territorio in cui viene individuato il sito per lo stoccaggio delle scorie nucleari, dal momento in cui iniziano i lavori devono sparire completamente la disoccupazione, i problemi ambientali, le opere non terminate e tutto il resto d'Italia dovrebbe contribuire a pagare per questo, puntando esclusivamente su procedure condivise, come si fa in altri Paesi, forse più civili del nostro. Questo è il motivo principale per cui mi oppongo: perché la Commissione non ha avuto il coraggio di chiedere una correzione del decreto, escludendo completamente l'ipotesi di imporre un deposito nucleare,

al quale non si opponevano la Provincia e la Regione; sapete tutti come è andata a finire: una rivolta popolare ha costretto il Governo a fare marcia indietro. Questo documento

tra i quali bisognerà scegliere un sito, e il Governo la tiene nel cassetto? Certo che la tiene nel cassetto, perché il 17 aprile c'è il *referendum* sulle trivelle e il Governo si guarderà bene dal rendere nota la scelta del sito.

nel cassetto. Perché questo? Perché nel momento in cui saranno resi noti i nomi dei potenziali siti, avremo tante rivolte locali di sindaci, di amministratori, del vescovo, del parroco, della Confindustria, della Coldiretti, i quali imporranno il ritiro delle località: una perché sismica, un'altra perché è la Sardegna, un'altra perché antropizzata. Se si volesse essere seri, come in tutta Europa,

come potenziali siti, e poi un termine entro il quale il sito viene accolto, altrimenti - ed è per questo che esprimo il mio dissenso - vi dico fin d'ora che questa è una pantomima,

parliamo di un tema un po' particolare: Poste italiane e uffici postali, perché credo ci sia la necessità da parte del Governo di intervenire immediatamente sulla chiusura degli uffici postali nel nostro Paese. La cosiddetta razionalizzazione degli uffici postali non sembra portare buoni frutti. Ora, non so se il metodo che è stato scelto, della concertazione e dell'ascolto degli amministratori locali interessati prima di operare scelte che incidono direttamente sul cittadino, adottato dall'ANCI e da Poste italiane stia dando buoni frutti, ma non sembrerebbe, perché sono accadute delle cose. Il Consiglio di Stato si è dovuto occupare della chiusura di presidi inutili ed inefficienti da parte di Poste italiane e della contrarietà da parte dei Comuni, tesa ad evitare disagi alla popolazione anziana residente. Nel caso in esame, un Comune pugliese aveva indicato alcune forme di contribuzione diretta all'ufficio periferico, pur di sostenerlo e farlo rimanere ovviamente il Consiglio di Stato reputa che con tali interventi si correrebbe il rischio di andare incontro a degli aiuti di Stato. Questo è un caso,

tratta ben 41 Comuni a cavallo tra le Province di Asti, Cuneo e Alessandria, interessate dalla decisione di far recapitare la posta a giorni alterni. Questa volta i giudici promettono decisioni veloci. Si tratterà di una causa pilota, perché i Comuni interessati a questa razionalizzazione sono 4.721, più della metà di tutti i Comuni italiani. Le dico inoltre che

nel mio territorio, in Abruzzo, soprattutto nell'entroterra della città di Vasto, che subisce queste stesse problematiche. Voglio ricordare che la direttiva europea afferma la garanzia del recapito postale per almeno cinque giorni a settimana e tale condizione è derogabile solo in presenza di circostanze o condizioni geografiche eccezionali. Quello che sta diventando eccezionale, in negativo, è la condizione degli abitanti. oltre metà dei Comuni italiani sono colpiti dalla cosiddetta razionalizzazione. Ora, chiedo con forza che chi governa trovi soluzioni soddisfacenti, evitando macchie di leopardo in Italia, ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato

La struttura di Secondigliano di Napoli è stata chiusa nel dicembre 2015, mentre quella di Castiglione delle Stiviere ha solo cambiato nome, trasformandosi da OPG in residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, in cui oggi sono ricoverate oltre 220 persone, ex internati, ora ricoverati, vorremmo poter dire a tutti gli effetti pazienti ospitati e curati, dalla stessa struttura in cui quelle persone sono state ristrette per molti lunghi anni. Altre 230 persone sono oggi ricoverate nelle REMS, quelle strutture che alcune Regioni hanno costruito e dove sono state quasi sempre semplicemente trasferite le persone ex internate negli OPG, alle quali viene assicurato un ambiente certamente più accogliente e meno degradato di quello in cui hanno vissuto per lunghi anni, ma alle quali viene ancora offerta una misura prevalentemente detentiva e non un vero e proprio percorso diagnostico-terapeutico-riabilitativo, in grado di favorire il loro recupero e l'inclusione sociale delle stesse. È grave la lentezza con la quale molte Regioni hanno dato attuazione alla legge n. 81 del 2014, pur con diverse situazioni: alcune Regioni si sono mosse più celermente, mentre altre sono molto indietro, tant'è vero che ben sei Regioni risultano inadempienti (Piemonte, Veneto, Toscana, Abruzzo, Calabria e Puglia). Queste sono state recentemente commissariate, come previsto dalla legge n. 81 del 2014 e come la Commissione sanità ha più volte sollecitato il Governo a fare.

purtroppo prevale ancora la logica custodiale: poca o nessuna possibilità di attività esterne alla struttura, guardie giurate armate, filo spinato, sbarre alle finestre. Anche la logica sanitaria, terapeutica e riabilitativa non sempre è adeguata. Riteniamo allora che il modo migliore per ricordare questo anniversario, fuori da ogni retorica e con uno spirito collaborativo,

e non necessariamente solo per un trasferimento nelle REMS - delle persone ancora internate negli OPG superstiti, così da chiuderli in via definitiva; definitiva; agire, nel rispetto delle prescrizioni della legge n. 81 del 2014, soprattutto per garantire che le misure alternative alla detenzione siano la norma e non l'eccezione (come purtroppo succede ancora spesso); spesso); procedere con urgenza ad adottare un atto che impedisca - o renda eccezionale - l'invio improprio delle persone in misura di sicurezza provvisoria in REMS, fenomeno che, come l'invio di detenuti dal carcere, sta ritardando la chiusura degli OPG (qualcuno si adopera a svuotare gli OPG, ma c'è qualcun altro che riempie i posti che restano vuoti); garantire, salvo casi eccezionali (che sappiamo possono sempre esistere) il rispetto della territorialità

all'indomani dei fatti di Bruxelles il presidente Renzi ha convocato il Comitato per la sicurezza, al quale ha partecipato anche il ministro Alfano.

In un primo *post* mette la foto di Putin e lo definisce un vero criminale che prova le proprie armi in Siria.

c'è chi beneficia dal terrorismo e questi sarebbero i regimi dittatoriali, che finanziano il terrorismo al fine di destabilizzare la situazione e continuare a rimanere al potere.

ci sarebbe da riflettere e la cosa è veramente molto grave. Se avessi saputo che questo Movimento, che doveva essere di critica, ma anche di miglioramento, avesse portato non solo a non migliorare le cose, ma addirittura a scavare, probabilmente non mi sarei mai candidata e non avrei fatto quello che poi ho fatto. Purtroppo, l'ho fatto. Il Movimento ha sempre più consensi, però insieme ad essi aumentano la disinformazione, la strumentalizzazione delle notizie e l'offuscamento dei fatti e dei dati. Ad esempio, questo Movimento si richiama sempre alle regole. Ma quali regole? Quelle che dicono loro e che poi non rispettano, quelle che interpretano diversamente a seconda che riguardino loro o altre persone.

Questore che appartiene a un Gruppo politico che spesso ha un atteggiamento molto esuberante in quest'Aula e che crea una